martedì sera è scomparso il senatore Sergio Zavoli. Giornalista e scrittore d'incredibile talento e brillante intelligenza, è stato tra i più vivaci e importanti narratori della nostra storia. Entrato in RAI giovanissimo, fu ideatore e conduttore di molte trasmissioni d'inchiesta e approfondimento. Il suo volto e la sua voce divennero per milioni di italiani la garanzia di un giornalismo di qualità, fatto di passione, ricerca instancabile della verità e rispetto. Aveva iniziato la sua esperienza in RAI dal giornalismo sportivo: indimenticabile il suo «Processo alla tappa» del Giro d'Italia, nel pieno degli anni '60, in cui riuscì a fondere sport e cultura, coinvolgendo nella sua trasmissione intellettuali del calibro di Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia. Seppe innovare, mostrando il lato umano della competizione, fatto di fatica, sacrificio, lavoro e lavoro di squadra.

presidente della RAI, dal 1980 al 1986, affrontò la sfida del superamento del monopolio della TV di Stato nella convinzione che il pluralismo e la concorrenza fossero un mezzo di promozione della crescita culturale e civile della società. Innumerevoli le sue pubblicazioni letterarie in cui il suo avvincente stile espressivo non usciva mai dal perimetro della fedele ricostruzione storica e biografica delle vite dei tanti personaggi che ci ha raccontato e dei fatti che ci ha spiegato. Far conoscere i fatti nella loro realtà, illustrarne ogni dinamica, ogni circostanza, ogni interesse e ogni finalità era per lui il modo migliore per toccare e risvegliare le coscienze, per portare tanto il lettore quanto il telespettatore a riflettere, a farsi domande, a non accettare mai passivamente le notizie. Eletto per la prima volta al Senato nel 2001 e poi per altre tre legislature, in ogni suo intervento seppe distinguersi per autorevolezza, competenza, serietà e grande rispetto per l'istituzione parlamentare. È stato motivo di grande dispiacere personale, di tutti i senatori e di tutta l'amministrazione non aver potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitaria tutt'oggi vigenti, la camera ardente qui in Senato per tributargli un ultimo saluto. Nel rinnovare, pertanto, la vicinanza mia di tutto il Senato ai familiari, ai parenti e agli amici del senatore Sergio Zavoli, invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

è stato ricordato dal Presidente, è stato un maestro del giornalismo e un pioniere, da quando Vittorio Veltroni identificò il suo talento di giovane ragazzo che faceva le radiocronache a Rimini per chiamarlo in RAI. È stato un pioniere che ha indicato la strada e

razionalità, semmai aridità, freddezza, mentre le poesie aprono uno squarcio nell'intimità delle persone. Eppure Sergio Zavoli era un poeta vero: ha scritto poesie meravigliose, ha scritto poesie meravigliose, che resteranno nel tempo. In tutto quello che ha fatto era un grande, riconosciuto tale dalle persone che lo hanno frequentato perché era autentico; quell'autenticità che non si può mascherare ma che emerge con forza nei contatti personali. Era così diverso dal tempo di oggi non soltanto per l'età, ma per caratteristiche. Siamo in un tempo in cui tutto è veloce, tutto è necessariamente superficiale perché la superficialità è figlia dell'accelerazione e della velocità. Il nostro è un tempo di grida, di aggressività. E invece Sergio Zavoli era l'opposto: era la forza della quiete, nel suo modo di parlare, nella pause di riflessione, nelle analisi; mai ostilità nei confronti degli avversari, mai aggressività nelle interviste straordinarie che faceva, interviste in cui la sua personalità era così forte da emergere in quella voce fuori campo che ha introdotto nella comunicazione italiana. Non c'era bisogno di farsi vedere: bastava la sua voce fuori campo - in quelle grandissime interviste che ricordiamo tutti - per riconoscere la sua autorevolezza. Zavoli era un uomo fuori dal tempo; era rimasto indietro. Colleghi, credo che la sua grandezza sia proprio in questo: non era indietro rispetto ai tempi di oggi, era più avanti; ci ha indicato semplicemente la strada che il Paese dovrebbe percorrere, con quei valori e con quei comportamenti che ci ha mostrato per tutta la vita. Continuerà a farlo dalla sua Rimini. In fondo sarà per sempre nella Rimini di «Amarcord», insieme al suo amico Fellini, ad indicarci la strada.

e c'è un verso di una sua poesia che voglio ricordare: «E mi riparo in ciò che accade». Cercare riparo nella realtà, nella vita: questa è stata la cifra del suo impegno. E ancora: «Far conoscere i fatti è già un modo di risvegliare le coscienze». E si capiscono allora tanti avvenimenti della vita di Sergio Zavoli. Si capisce allora perché nel 1962 abbia portato la televisione, per la prima volta, all'interno di un istituto psichiatrico a Gorizia, dal dottor Basaglia. Conoscere e risvegliare le coscienze: è questo che gli fa fare le interviste più belle, con la sua voce che testimoniava la partecipazione emotiva che lo portava a contatto a rivolgere anche le domande più scottanti. Detestava l'informazione ammiccante, enfatica, sin dalla sua prima grande innovazione televisiva che fu il «Processo alla tappa»: un viaggio nelle storie, nelle emozioni, nella vita dei gregari del Giro d'Italia,

Tutto questo è Zavoli giornalista, ma la stessa identica passione, impegno, intelligenza e ironia hanno caratterizzato l'attività del senatore Sergio Zavoli, che ha lasciato il segno in quest'Aula, un segno garbato ma potente. Sergio Zavoli ci mancherà, ma mancherà soprattutto l'idea etica dell'informazione e della partecipazione politica, così lontana dal panorama sguaiato di questo nuovo millennio. Grazie, grazie per sempre Sergio Zavoli!

Per me bambino il primo ricordo di Zavoli è il presidente della RAI Sergio Zavoli: sembrava una frase tutta attaccata nei TG di allora. Poi l'ho scoperto nella libreria di casa, autore di alcuni volumi che evidentemente erano importanti tanto da avere un posto significativo. Poi abbiamo imparato a conoscerlo - come veniva ricordato da ultimo anche dal collega Bressa - come il grande narratore di storie, non soltanto delle storie epiche. Intervistava la maglia nera del Giro d'Italia e il "cannibale" Merckx; era cioè capace di raccontare l'umanità dentro la battaglia sportiva. Poi, ancora, c'è l'amicizia con Federico Fellini, con un'immagine bellissima (non la conoscevo, l'ho imparata in queste ore rileggendola sui giornali), in cui Zavoli dice che loro da piccoli sognavano a colori. È un'immagine fantastica: gli altri sognavano in bianco e nero e loro sognavano a colori. È bello nella tragedia che questo 2020, anno del centenario di Federico Fellini, li riavvicini come saranno vicini per sempre nella loro Rimini, terra alla quale era attaccato. Quando scoprì che nel mio sangue c'è un quarto di sangue romagnolo cambiò sguardo verso di me. Da allora mi salutava dicendo «auguri romagnoli». Aveva accettato la sfida del giornalismo e della qualità, ma poi aveva accettato la sfida della politica. Ha fatto bene il ministro Franceschini a ricordare Vittorio Veltroni, e credo sia altrettanto giusto ricordare come il suo impegno nella cosa pubblica sia arrivato sulla base di una richiesta di Walter Veltroni, cui va il nostro ringraziamento. Un impegno che lo ha portato ad assumere posizioni rilevanti anche all'interno della Commissione di vigilanza RAI e non soltanto nell'Aula del Senato, e che lo ha portato (perlomeno per quello che mi riguarda) a vivere alcune pagine che resteranno per sempre nella mia memoria personale, Dopo lunghe notti di discussione parlamentare - se lo ricorderanno anche gli amici che allora stavano all'opposizione facendo ostruzionismo il nostro Gruppo lo vedeva praticamente sempre presente in Aula e noi per primi, dai banchi del Governo, ci preoccupavamo di Sergio e della sua resistenza. dopo un passaggio particolare, il 14 ottobre del 2015, lui si presentò in Aula dopo una notte di discussioni e dopo tanto ostruzionismo, giustamente la differenza tra i tempi - è che gli SMS passano, ma i bigliettini di carta rimangono. Dai banchi del Governo gli mandai un bigliettino per ringraziarlo e dirgli quanto gli fossimo debitori per la sua dedizione, indipendentemente dal voto che aveva espresso in quella vicenda della riforma. Lui mi ha scritto delle parole che resteranno con me per sempre: «Caro Presidente, alla mia età, se non faccio più il mio dovere posso solo dimettermi da me stesso. Grazie per quello che mi scrivi. Auguri a te forti romagnoli». Sergio Zavoli è stato il giornalista che per definizione è il contrario delle *fake news*. Era l'anti-*fake news* per definizione. Era l'uomo che cercava la verità. E quanto sarebbe bello che la Commissione parlamentare che dedicheremo alle *fake news* nelle prossime settimane e nei prossimi mesi lo ricordasse dedicandogli spiritualmente i lavori. Si dedicano le stanze, si dedicano le Aule; sarebbe bello che dedicassimo i lavori di quella Commissione esattamente a un maestro come Zavoli. Quanto sarebbe bello per chi fa politica che nell'Aula in cui ascoltiamo il Primo Ministro e tutti i Ministri ci ricordassimo di qualche maestro. Sì, perché il latino ci insegna che «maestro» vale più di «ministro»: maestro viene da *magis,* mentre ministro viene da *minus*. Se saremo in grado, anche nel prosieguo della legislatura, di ricordare un maestro quale Sergio Zavoli, credo che avremo fatto un passo importante nella strada di testimoniare la fedeltà alla memoria di un uomo che è stato un secolo di civiltà per tutti noi.

Sì, colleghe e colleghi, Sergio Zavoli ha scritto le pagine più belle del giornalismo radiotelevisivo che hanno fatto la storia del nostro Paese e del servizio pubblico del nostro Paese. come scrittore, politico, amico di Federico Fellini, socialista di Dio, sì, senatore, Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, presidente RAI, direttore di giornali, ma consentitemi, in questa occasione, con grande umiltà, di provare a trasmettervi le emozioni che provo oggi nel tratteggiare una figura così importante per il giornalismo del nostro Paese.

alla difesa delle conquiste operaie contro l'avventurismo brigatista, per fare solo qualche esempio [...] dai giorni di Reggio Calabria a quelli di Reggio Emilia, dagli scenari dello stragismo a quelli degli anni di piombo, fino al caso Moro, e poi a Ruffilli, a D'Antona Un vero intellettuale, protagonista del giornalismo civile al servizio del suo Paese. Per lui la parola era sacra, aveva un senso altissimo delle istituzioni, una grande umanità. Lo ricorderemo per il suo «Processo alla tappa», che insegnò un modo nuovo di raccontare lo *sport*, per la sua «La notte della Repubblica», per il documentario radiofonico - che oggi noi chiameremmo

che entrasse in vigore la legge n. 180 che aboliva i manicomi. Mi devo fermare qui, pur sapendo di fargli un torto, ma quello che mi preme sottolineare in questo momento è la qualità della sua narrazione: cinematografica. Rapito dalla bellezza, era meticoloso, pignolo nel suo lavoro, tutto doveva essere perfetto, in radio come in Ho avuto il privilegio di imparare - non so fino a che punto ci sia riuscito - a fare radio con chi aveva lavorato con lui. Per fare TV - si diceva un tempo - bisognava saper fare radio, bisognava leggere senza inflessione dialettale mi dicevano i tecnici, e dopo pranzo mi costringevano a leggere ad alta voce un articolo suggerendomi la pausa, il timbro di voce, la freddezza nel racconto. Questa era la RAI: straordinarie professionalità e orgoglio di lavorare per il servizio pubblico. Tutti ci ricordiamo la voce di Sergio Zavoli, eccome se sapeva scrivere: di luce delle sue interviste e se c'erano silenzi non erano tempi morti, facevano parte del racconto. La sua non era una TV urlata, ma profonda, d'inchiesta, di approfondimento. Si dice che il giornalismo di Zavoli non cercasse lo *scoop*,

Musica, immagini, suoni, voce narrante, testimonianze; asciutto, essenziale, profondo, le sue inchieste prendevano forma nelle sale di montaggio. Quando c'era l'intervistato in primo piano, le sue domande erano con la voce fuori campo. Altri tempi, altro stile. Era un cronista perché era curioso e le sue inchieste erano avvincenti perché non aveva una tesi precostituita, che non significava non avere un punto di vista. Non credo che ci possano essere eredi, non esistono eredi, certo nella RAI degli anni di Sergio Zavoli sono cresciuti giornalisti con la G maiuscola, le generazioni successive sono andate oltre quel modo di fare giornalismo: meglio? Peggio? Io so che quando finivo di vedere o di ascoltare un'inchiesta di Sergio Zavoli, dicevo: canone per il servizio pubblico. La qualità della democrazia dipende dalla qualità e dalla libertà del giornalismo. Nei tempi delle notti della Repubblica c'era lui, Sergio Zavoli, e tanti altri come lui che hanno acceso i riflettori e fatto crescere la coscienza civile. Ciao, direttore.

Sergio Zavoli era un intellettuale, un giornalista, Presidente di una grande azienda pubblica, scrittore, poeta. È stato anche senatore per quattro legislature, fino al 2018. A me capita oggi di ricordarlo proprio dal banco che è stato suo fino all'ultimo giorno della legislatura passata. Molti di noi lo hanno conosciuto personalmente e qualcuno di noi gli è stato amico, ma tutti lo abbiamo ammirato e non solo per la sua finezza ed equilibrio politico, ma anche per il suo valore culturale e intellettuale. Rare volte mi è capitato di incontrare in Parlamento personalità, giganti come ha detto poco fa il ministro Franceschini, con un'uguale passione politica, profondità culturale e sensibilità umana ed è difficile ricordarlo senza provare una grande commozione. Gli sono stato vicino nei tanti anni passati insieme al Senato, anni politicamente difficili ma nei quali c'era ancora chi, come lui, intendeva la battaglia politica non solo come tattica per il primato, ma anche come battaglia delle idee. La mia amicizia con lui è iniziata molto prima del suo e del mio ingresso in Senato, perché ci siamo conosciuti negli anni Settanta quando tutti e due eravamo molto più giovani, nel tempo in cui Sergio Zavoli arricchiva la vita sociale e culturale del nostro Paese con il suo straordinario lavoro di giornalista e direttore, di autore di inchieste esemplari per la completezza dell'informazione e per l'assenza sempre di qualsiasi pregiudizio. È l'insieme di questi ricordi che mi fa dire che Sergio Zavoli era un uomo limpido e un senatore leale: leale con la sua Romagna, con la sua Rimini, che ha amato sino alla fine; leale con gli amici della giovinezza, primo tra tutti Federico Fellini; leale con i suoi colleghi senatori. Io ricordo molto bene la tenerezza con cui si rivolgeva alle senatrici sue amiche, Anna Finocchiaro, Mara Valdinosi, Roberta Pinotti e Valeria Fedeli. però era leale e limpido nell'orgoglio di essere un senatore del Partito Democratico. Uomo di Sinistra, testimone dei valori della democrazia parlamentare e del ruolo che i grandi partiti popolari hanno avuto nella storia della Repubblica, Sergio Zavoli sapeva leggere molto bene la società italiana nelle sue virtù e nel suo degrado. La vedeva ingrigita - lo cito nel troppo tempo concesso alla dimenticanza, all'ambiguità, all'arrendevolezza e persino alla menzogna. Ma neanche davanti ad un'analisi così impietosa Sergio Zavoli si è mai arreso, perché era un vecchio riformista e - lo cito ancora con una naturale inclinazione persino verso una temerarietà ben governata. Ed è per questa sua natura di uomo con la testa rivolta al futuro Sergio Zavoli, parlando di se stesso ma rivolgendosi ai colleghi senatori, diceva (sentite): «Se avessi una qualche abilità persuasiva, immodestamente vi inviterei, presenti ed assenti, a credere che si cresce grazie ai problemi che si è costretti a risolvere, che è bene risolvere e che è urgente risolvere, nella convinzione che si racchiude in una parola: insieme». Sono parole molto importanti anche per noi, ci riguardano da vicino e sono di un'attualità impressionante. Anche oggi, la strada più diretta per far uscire l'Italia dalla grave crisi che sta attraversando è la stessa che anni fa ci indicava Zavoli e che si racchiude in una parola: insieme. Dicendo «insieme», Zavoli voleva dire «basta con l'individualismo, basta con le divisioni e le sottodivisioni, basta con l'uso strumentale del Parlamento». Oggi probabilmente a Sergio sarebbe piaciuto essere ricordato in Senato per la sua vita così piena e così avventurosa; intanto per il suo lavoro di giornalista sportivo, perché è lì che ha appreso il mestiere del grande inviato, imparando quanto nelle vicende umane siano importanti le singole persone e anche gli ultimi e quanto valgano la fatica e i sacrifici di chi si mette in gioco in quelle gare dove, come al «Giro d'Italia», non è ammesso che qualcuno si risparmi. Lo sport, se non è leale, non è sport e Zavoli ha insegnato all'Italia quanto per tutti noi può valere vivere osservando un codice deontologico. Ma gli sarebbe piaciuto anche essere ricordato per le sue grandi inchieste giornalistiche, per la sua testimonianza sui pericoli eversivi corsi dalla nostra democrazia e sulla vittoria della democrazia e dei valori della Repubblica. essere ricordato come uomo di sinistra e senatore del Partito Democratico, di un partito in cui il dibattito interno è sempre stato vivace e libero, ma in cui l'unità politica resta un valore. Gli sarebbe piaciuto essere ricordato per il suo lavoro in Senato, dove la maggioranza e l'opposizione l'hanno sempre ascoltato nel più assoluto silenzio, segno dell'interesse per quel che diceva, ma anche di rispetto pieno per la sua persona. Infine, gli sarebbe piaciuto essere ricordato per le sue poesie, nelle quali riversava la sua umanità e la sua sensibilità; poesie dalle quali traspariva il mistero di un uomo pubblico che si confronta con i propri struggimenti personali. Anche per me, come per tutti quelli che mi hanno preceduto, fra i tanti ricordi che hanno affollato la mia mente quando ho saputo della sua scomparsa, il ricordo più forte è quello della sua voce; una voce che abbiamo sentito alla radio, alla televisione, una voce che abbiamo ascoltato con attenzione nell'Aula del Senato; una voce bellissima, fascinosa, calda, profonda e chiara, che esprimeva insieme i suoi pensieri, ma anche tanto della sua personalità e dei suoi sentimenti; una voce che mi colpiva ogni volta che parlavo con lui negli angoli tranquilli del Senato o lo sentivo al telefono o quando mi chiedeva di andare a mangiare insieme, perché - diceva - si parla meglio. Ho ancora nelle orecchie la voce di Sergio Zavoli ed è proprio il suono della sua voce che me lo fa sentire ancora vivo.

che ha segnato, con uno stile e un linguaggio tutto suo, un'intera epoca. È stata l'unica personalità nella storia della RAI ad aver ricoperto tutti i ruoli: è stato giornalista (e che giornalista!), autore di inchieste e programmi, dal «Processo alla tappa» fino a «La notte della Repubblica», pietre miliari nella storia del giornalismo italiano. Ma fu anche direttore del GR1, vicedirettore del TG1, Presidente della RAI e ha presieduto la Commissione parlamentare per l'indirizzo Ruoli svolti in un periodo di grandi trasformazioni e vitalità del panorama radiotelevisivo, che ha ricoperto sempre con grandissimo senso delle istituzioni. Non è mai stato un giornalista da *scoop* o da notizie «mordi e fuggi», ma ha sempre usato la notizia per comprendere, analizzare, indurre alla riflessione. Come ha ben detto ieri Aldo Grasso in un suo ricordo: «Zavoli ha dato alla TV il diritto di riflettere». Aveva uno stile intelligente e mai superficiale, e la compassione umana, merce rara in chi fa il suo mestiere, era un suo tratto identitario, che si trattasse di suore di clausura, di ciclisti e financo di terroristi. Ma in questi anni di inutile e dannoso tentativo di mistificare la storia, è stato detto che Sergio Zavoli era un socialista; certamente, «Socialista di Dio» si autodefiniva, come recita il titolo di un bel suo libro di memorie. Ma nessuno ha detto, anche nelle commosse ricostruzioni, Sergio Zavoli negli anni Ottanta è stato membro dell'assemblea del Partito Socialista Italiano: la tanta vituperata e impropriamente aggettivata assemblea «dei nani e delle ballerine», a riprova invece dello sforzo che, all'insegna della qualità, il nuovo corso craxiano intese imprimere alla politica italiana attraverso l'apertura del partito alle migliori intelligenze del panorama culturale, artistico e intellettuale di un'Italia che aggrediva il futuro. Mi è capitato, in questi anni di esperienza parlamentare, di incontrare e colloquiare con Sergio Zavoli. Avevamo compiuto scelte diverse, ma non è mai mancato il rispetto e, ancora di più, non è mai mancato il sentimento forte di appartenere a una stessa comunità.

Signor Presidente, non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Sergio Zavoli, ma ho dei ricordi: il mio primo ricordo è TV7, un appuntamento imperdibile di approfondimento; ero solo una bambina, ma ne ricordo perfettamente i servizi. Poi ho avuto modo di conoscere, attraverso questa voce inconfondibile e profonda - come lo era lui -, molti suoi interventi. interventi. Indimenticabile «La notte della Repubblica»: cinquanta ore di testimonianze e di approfondimenti su una delle pagine più buie della storia della nostra Repubblica.

Parlando del servizio pubblico, diceva: «Uno straordinario mezzo di promozione della crescita culturale e civile della società», quindi fondato sulla verità. E un'altra cosa fondamentale: «Far conoscere i fatti è già un modo di risvegliare le coscienze». Quindi l'insegnamento che la consapevolezza è la base per prendere le decisioni. Era un intellettuale vero, figlio del suo tempo, dico io. Nato nel 1923, aveva quel rigore morale ed intellettuale, quell'impegno e quel senso civico che dovevano durare tutta la vita. Era come una *conditio sine qua non*: così bisognava essere cittadini, da qualunque ruolo, bisognava portare avanti un impegno sociale con tanto senso civico. Disse una frase che ancora una volta ci coinvolge tutti e la pronunciò proprio in quest'Aula: «Questo mondo ha bisogno di essere cambiato e ci chiede di farlo», cioè ognuno deve fare la sua parte. Questa direi che è un'eredità molto, molto consistente. Zavoli ci ha dato strumenti per capire la verità. Ha avuto una grande attenzione ai deboli perché la consapevolezza, sia da giornalista ma anche poi da politico, significava conoscere anche chi era meno visibile, perché erano le vite di persone. Una frase incredibile mi ha sorpreso, ma era in continuità e in coerenza con quello che è stato: «Non vorrei andarmene senza essere presente al congedo. Dopo l'evento della mia nascita, vorrei non perdermi quello, conclusivo, del congedo», cioè essere sempre lucido, vivere ogni piccolo istante, capire capire il mistero della vita, esserci, quasi a doverlo testimoniare ancora, anche se è l'ultimo atto. Incredibile. Penso che un personaggio di questa levatura abbia onorato il nostro Paese ha fatto da intellettuale raffinato, ma ironico, sempre spinto da questo spirito di servizio. Ritengo che l'Assemblea tutta e il Paese perdano un figlio importante, che è stato testimone di un secolo, ma è stato anche protagonista dell'esser testimone: è sempre stato in prima persona a governare la sua vita e ad orientare anche quella degli altri, ma nel senso della verità. Penso sia stato un grande maestro e per questo onoriamo la sua morte con tanto rispetto e cogliendo gli insegnamenti

Signor Presidente, onorevoli senatori, la scomparsa di Sergio Zavoli ci addolora profondamente. Da quest'Assemblea, che lo ha accolto per diciassette anni, giungano i sentimenti di vicinanza e cordoglio del MoVimento 5 Stelle ai suoi familiari e ai suoi colleghi del Partito Democratico. Zavoli è stato un protagonista del giornalismo italiano e della vita civile e culturale della nostra storia recente. Con lui scompare una grande voce di libertà, uno dei più importanti giornalisti dell'Italia del Dopoguerra, un punto di riferimento ideale e morale nel mondo dell'informazione e della televisione. Zavoli era personalità di grande rigore intellettuale, che ha costantemente interpretato, al servizio del pluralismo e della libertà dell'informazione, i valori della democrazia, testimoniati da una convinta adesione ai valori della nostra Costituzione. In anni in cui ogni tipo di informazione e conoscenza correvano correvano il rischio di essere assoggettati alla logica del mercato e schiacciati nella morsa della politica, da giornalista radiotelevisivo Zavoli ha praticato la professione con sensibilità, intelligenza, passione e rigoroso rispetto per la realtà dei fatti raccontati. Lo ha fatto come pochi, da giovane cronista radiofonico approdato nella Roma del Secondo dopoguerra. Egli ha garantito ad altri - a tutti - di farlo anche quando della RAI è diventato Presidente socialista in anni complicati, da orgoglioso e geloso custode della missione autentica del nostro servizio pubblico radiotelevisivo;

proprio per questo, lui, meglio di tutti, quel tempo voleva scrutarlo, indagarlo e soprattutto capirlo. Lo ha fatto con inchieste che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo italiano:

quando, da esempio raro per un politico, amava intrattenersi con i cronisti più per farli parlare e conoscere che lasciarsi intervistare. Per Zavoli era una necessità capire, così com'era una necessità civile e morale raccontare; insomma il cuore e l'essenza del giornalismo che Zavoli è riuscito a coniugare e dispiegare come pochi altri nel nostro Paese. Era anche convinto che la televisione potesse essere uno strumento per cambiare in meglio questa società, così come credeva fermamente che il giornalismo dovesse sforzarsi di preservare in purezza le sue radici, a partire proprio dal servizio pubblico che doveva rivendicare ogni ogni giorno, diceva, l'autonomia della propria missione culturale informativa. Per questo la sua scomparsa non solo ci addolora per il vuoto che lascia ma ci interroga su temi importanti del nostro tempo, sulla qualità del lavoro giornalistico e sul rispetto dei diritti dei lavoratori dell'informazione, su un'informazione libera e indipendente che ci permetta di diventare cittadini consapevoli dei nostri diritti e non sudditi. Questa è l'eredità che ci lascia Sergio Zavoli. L'amore per l'Italia e la conoscenza della storia nazionale hanno ispirato la sua opera di giornalista, di scrittore, di poeta, così come le sue indagini nel corpo vivo della realtà italiana. Il giornalismo era per lui la chiave per aprire la porta alla conoscenza del Paese, per scendere nella sua più intima essenza per sondarne e indagarne bellezza e complessità, pagine straordinarie di un percorso umano e professionale che hanno scolpito in maniera indelebile il nostro immaginario di spettatori, lasciando nel contempo una preziosa traccia e preziosi semi nella nostra coscienza di cittadini. Questo è il mio, il nostro saluto a Sergio Zavoli, un uomo che ho avuto il privilegio di conoscere, di sfiorare prima, poi apprezzare e infine vivere professionalmente in questo palazzo. Certo, Sergio, resta il rimpianto di quelle pagine di romanzo non lette insieme mentre si formavano, ma che in fondo potrai sfogliare nel luogo di pace e serenità, ovunque esso sia, che ti sei scelto e che meriti. Il mio saluto fondamentalmente vuole essere anche un augurio, soprattutto a quelle nuove generazioni che si affacciano nel mondo del giornalismo. L'augurio è di seguire l'esempio di Sergio, di quei pochi buoni maestri, ormai sempre più rari, che ogni giorno cercano la chiave di conoscenza che possa possa spalancare finestre e stanze del nostro vissuto per lasciar entrare la luce della consapevolezza laddove c'è il buio dell'abbandono e dell'indifferenza, un lavoro che lui ha svolto con grande onestà intellettuale, senso delle istituzioni ed intensa partecipazione umana, come ha fatto oggi notare un autorevole commentatore. Di questo siamo grati a Sergio Zavoli, simbolo ed alfiere del servizio pubblico che noi vorremmo e per questo lo ricorderemo sempre con sincero affetto e grandissima ammirazione.

Presidente, la ringrazio moltissimo per questa possibilità.

perché, almeno per me, il senatore Sergio Zavoli è ancora seduto al suo posto, con i suoi occhi scintillanti, il suo acume, la sua intelligenza, e il suo sguardo di profonda umanità. Credo che, se noi sentiremo, come lo sento io, quello sguardo e, quindi, anche

così Sergio Zavoli definiva l'importanza e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo. Per il suo contributo da protagonista la cultura e alla vita democratica del nostro Paese

Per tutta la vita al centro degli eventi determinanti della storia italiana, Zavoli ha saputo affrontare i temi più complicati perché fossero compresi dai cittadini comuni, parlando alla radio e alla televisione con il linguaggio di un giornalismo spontaneo e attento alla persona. Il suo stile di racconto, dalle cronache ricordate del Giro d'Italia a "La notte della Repubblica", è diventato patrimonio della società e del costume. La sua capacità più grande è stata quella di porre, e porsi, sempre domande giuste, con parole semplici. Uomo di cultura raffinata, non cercava il consenso, ma lavorava piuttosto per lasciare un dubbio, approfondire, aprire nuovi spazi di dialogo. La sua presidenza RAI e quella della Commissione per la vigilanza RAI sono state un esempio di pluralismo e rispetto delle regole delle istituzioni. La sua voce equilibrata, autorevole e profonda, il timbro di un'Italia la cui eredità deve renderci orgogliosi del nostro passato e responsabili del nostro presente e del nostro futuro.

Oggi, come diceva Sergio Zavoli, abbiamo bisogno di capire, perché viviamo un tempo che, per molti versi, non ci piace. Senatore Barachini, questa mi sembra una bella iniziativa, che appoggio con piacere. Io mi auguro, come diceva prima il senatore Renzi, che in quell'Aula risuonino anche tutte le sue iniziative. *(Applausi)*.

il "Processo alla tappa", così come si è inventato la "Notte della Repubblica". Passava da un argomento all'altro, con il gusto del giornalista che sa approfondire ma che sa anche inventare. Credo che egli sia stato l'ultimo dei giornalisti

alla Camera dei deputati, ha la finalità, in una situazione ovviamente eccezionale, di dare piena attuazione al principio costituzionale dell'accesso paritario alle cariche elettive, anche nello svolgimento delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia, fissate per il 20 settembre prossimo. dire subito che si tratta di un provvedimento di grande valore istituzionale e politico, dal momento che in gioco ci sono non solo diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine pugliesi, ma la stessa qualità della democrazia e, in fondo, l'idea stessa di democrazia che abbiamo tutti. Anche per questo voglio rivolgere un ringraziamento a tutte le forze politiche e soprattutto a quelle di opposizione,

L'esigenza di questo provvedimento di urgenza, come tutti sappiamo, deriva da un fatto specifico, francamente poco opinabile, sia sul piano della realtà, sia su quello giuridico e, infine, credo di poterlo dire, anche dal punto di vista politico. Prima però di arrivare a questo, vorrei fare un passo indietro: il quadro normativo nel quale il provvedimento in esame si colloca è definito da una legge, che il Parlamento ha approvato definitivamente nel 2016, che a sua volta ha modificato la legge n.165 del 2 luglio 2004, con la quale si era inteso dare attuazione all'articolo 122 della Costituzione, norma che attribuisce alla legge ordinaria il compito di definire i principi fondamentali a cui devono attenersi i sistemi elettorali, anche regionali. Proprio grazie alle modifiche introdotte nella passata legislatura, quella legge, alle disposizioni generali sulla promozione della parità tra i sessi, unisce oggi anche alcune disposizioni specifiche, con l'obiettivo di prevedere meccanismi di tutela del genere meno rappresentato, tarandoli sui diversi sistemi elettorali. Tra questi, per stare soltanto ai sistemi con voto di preferenza, vennero introdotti due meccanismi: una presenza nelle liste elettorali di una quota minima del 40 per cento del genere meno rappresentato e la possibilità di esprimere la doppia preferenza a candidati di un genere diverso, con la conseguenza, in caso di violazione, della nullità della seconda preferenza espressa. Senza entrare nel merito di un dibattito che il Parlamento affrontò pochi anni fa, voglio però ricordare il contesto nel quale maturava quella legge: da una parte ci sono le riforme costituzionali degli anni 2000, come la riforma dell'articolo 51 della Costituzione, approvata nel 2003, che dispone che i cittadini hanno il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza alle assemblee elettive e prevede che la Repubblica promuova «con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne». poi la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, del 2001, per cui la normativa regionale deve intervenire per rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono «la piena parità degli uomini e delle donne» e promuovere «la parità di accesso tra donne e uomini» a tutte le cariche elettive. Infine c'è il già richiamato articolo 122 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni il potere di legiferare in materia di sistema elettorale delle assemblee elettive regionali, riservando tuttavia allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali. Da questo rinnovato quadro costituzionale nascono poi le numerose leggi regionali, che in questi anni hanno introdotto disposizioni sulla composizione di genere delle liste e sulla cosiddetta doppia preferenza di genere. Tra queste ricordo solo la prima, adottata nel 2009 dalla Regione Campania, un modello poi seguito dalle altre Regioni. Su questa legge, la Corte costituzionale si espresse con la sentenza n. 4 del 2010, che la dichiarò in linea con i principi ispiratori degli articoli 51 e 117 della Costituzione, in quanto entrambi espressione del principio di uguaglianza sostanziale contenuto all'articolo 3. quella sentenza cambiò il corso della storia su questo fronte. Ho voluto ricordare brevemente il quadro normativo e la storia di questi ultimi anni, perché fanno capire quanto difficile sia oggi tollerare ancora ritardi, dilazioni o, peggio, ipocrisie sul principio delle pari opportunità per le cariche elettive, che ormai da tempo è parte fondante dell'ordinamento nazionale e dell'immagine condivisa della nostra democrazia. Ora, il decreto-legge che stiamo esaminando al primo articolo fissa un principio del quale vi chiedo di considerare la rilevanza e cioè il mancato recepimento nella legislazione regionale dei princìpi ricordati in materia di sistemi elettorali costituisce uno dei presupposti per l'attivazione del potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, disciplinato da successiva legge di attuazione. Il secondo comma contiene disposizioni specifiche da applicare nella Regione Puglia in occasione delle elezioni del nuovo Consiglio regionale previsto per settembre 2020. In particolare, viene stabilito

le quali - lo sottolineo - sono assunte per assicurare il pieno esercizio dei diritti politici dei cittadini pugliesi per garantire l'unità giuridica della Repubblica e il rispetto dei princìpi fondamentali della nostra Carta costituzionale Le disposizioni di cui discutiamo sono le seguenti: la prima prevede che ciascun elettore potrà esprimere due voti di preferenza, una delle quali riservata necessariamente a un candidato di sesso diverso dall'altro; la seconda è che, nel caso in cui vengano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, la seconda sarà annullata; infine, sempre all'articolo 1, per dare piena e veloce attuazione alle norme precedenti, la prefetta di Bari viene nominata commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti richiesti per l'attuazione del decreto-legge e di verificare insieme la compatibilità delle disposizioni regionali con le nuove introdotte appunto dal presente decreto-legge relative alla doppia preferenza; i restanti due articoli contengono clausole d'invarianza finanziaria e disposizioni per l'entrata in vigore del decreto-legge. È chiaro allora, colleghi, che l'ambito d'intervento del decreto-legge è stato prodotto dal mancato adeguamento del sistema elettorale della Regione Puglia ai principi già introdotti fin dalla legge n. 165 del 2004 in materia di parità d'accesso alle cariche elettive. Mi rendo pienamente conto della delicatezza dell'ambito dell'intervento, relativo al sistema elettorale di una Regione, nel quale sarebbe rischioso creare precedenti attraverso un utilizzo poco cauto del potere sostitutivo pure messo a disposizione dalla Costituzione. Mi rendo conto di tutto questo, ossia del profilo non solo di legittimità, ma anche di opportunità: eppure, colleghi senatori, credo di poter valutare obiettivamente il dato di realtà di quanto è successo nelle scorse settimane e dei limiti che quest'intervento legislativo rispetta. Dovrebbe essere chiaro a ciascuno di noi che i presupposti di fatto e di diritto ricadono nel solco di quanto imposto appunto dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, che detta le norme attuative dell'articolo 120, comma, della Costituzione, a partire dall'esigenza di assegnare all'ente coinvolto - in questo caso, la Regione Puglia - un termine congruo entro il quale adottare provvedimenti dovuti o necessari relativamente al mancato adempimento degli obblighi previsti. Le date sono gli atti formali che, in questo caso, valgono più di molte parole a dire che appunto quel criterio di congruità è stato pienamente rispettato: dopo tutti i richiami informali, la lettera del ministro Boccia, con l'invito ad adeguarsi, reca la data del 5 giugno; stesso mese arriva l'informativa del ministro Boccia in Consiglio dei ministri, che segnala l'inadempienza; del 3 luglio è la nota ulteriore del presidente Conte, con l'invito a decidere con la massima urgenza; il 23 arriva la diffida formale con invito a provvedere entro il giorno 28, prospettando l'ipotesi di un decreto-legge; del 31 luglio la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri in rappresentanza della Puglia. La scansione delle date evidenzia come l'intervento del Governo sia stato reso necessario dalla prolungata inerzia del Consiglio regionale pugliese, cosa che semplicemente è nei fatti, ma soprattutto dimostra che sia stato concesso tempo all'Assemblea regionale per adeguarsi alla normativa nazionale e che sia stato congruo, soprattutto tenendo conto delle imminenti scadenze elettorali del 20 e 21 settembre prossimi. Un'ulteriore considerazione va fatta da ultimo in merito alla proporzionalità dell'intervento, condizione anche questa imposta dalla legge di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. La legge elettorale della Regione Puglia presenta un sistema proporzionale con preferenza: di conseguenza, l'intervento del Governo non poteva che orientarsi nella selezione tra diversi meccanismi previsti dalla legge del 2016, per promuovere parità di accesso alle cariche elettive, verso il modello della doppia preferenza, basata appunto sul genere. Anche su questo terreno, dunque, vi sono stati piena consapevolezza e rispetto da parte del Governo dei limiti che un siffatto intervento era tenuto ovviamente a rispettare. Proprio considerati gli elementi di cautela con cui si è operato nelle condizioni date, consentitemi allora una considerazione dal significato più politico per sottolineare l'importanza di un intervento che, per la prima volta, attiva i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione per affermare l'equilibrio di genere nella rappresentanza delle istituzioni. Molti lo hanno considerato un intervento sostitutivo di notevole portata; alcuni l'hanno considerato eccessivo; tutti - credo saremo d'accordo su questo - lo consideriamo un intervento che avremmo preferito non fare.

Dico soltanto che, se si usa questo potere di intervento per garantire parità tra donne e uomini, non si compie alcun abuso di potere, non si viola il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, non si sta restringendo la sfera dei diritti, ma al contrario la si sta semplicemente ampliando. Lo Stato sta semplicemente adempiendo al ruolo di protezione della sfera dei diritti, che devono essere tutelati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Il compito principale della nostra democrazia è proprio quello di far avanzare i diritti di tutti i cittadini in maniera uniforme; è questo il senso pieno dell'articolo 3 della nostra Costituzione che, nella piena collaborazione reciproca tra Stato, Regioni, Comuni ed enti territoriali, tutti devono perseguire. n. 216 del 2013, in materia di parità di genere nei Consigli regionali, venivano soprattutto dalla considerazione, ampiamente condivisa - dati alla mano - e dalla necessità di un intervento a livello regionale. Dopo quattro anni, quei numeri non sono cambiati molto: secondo i dati del febbraio 2020, la presenza delle donne nei Consigli regionali in media non arriva

L'obiettivo di superare tale squilibrio ci riguarda tutte e tutti, a prescindere dalla forza politica di appartenenza. È una di quelle sfide che impongono - credo - lo sforzo di lasciare un passo indietro le appartenenze agli schieramenti per far fare un passo in avanti all'interesse generale che tutti noi rappresentiamo. Lo abbiamo fatto già molte volte in passato; abbiamo più volte saputo trovare convergenze ampiamente maggioritarie proprio sul tema dei diritti delle donne e delle pari opportunità per tutte e tutti, a partire dalla convinta condivisione delle richiamate riforme costituzionali. Oggi con questo provvedimento abbiamo l'occasione di lanciare al Paese un ulteriore messaggio di coesione dinnanzi alla tutela e alla promozione dei diritti indiscussi e indiscutibili di ciascuno di noi. Chiedo a tutta l'Assemblea di farlo insieme ancora una

La materia apparentemente non sembra un granché: è tra quelli che possono essere definiti "decretini", che non è una parolaccia, ma si riferisce alla dimensione del decreto. Così probabilmente non è per il Governo che, invece, ha usato toni esaltanti nei confronti del provvedimento. Il presidente Conte, infatti, ha proclamato che con questo imperativo morale, politico e giuridico è stata scritta una pagina della storia italiana dei diritti politici. Il ministro Boccia - che saluto - ha dichiarato, invece, che la doppia preferenza appartiene alla categoria dei diritti universali. Il ministro Provenzano, invece, ha stabilito che si è trattato di un passo avanti nella lotta alle disuguaglianze. Nei corridoi il decreto non è stato considerato in questa maniera; lo considerano un "decretino". Lo chiamano in maniera impropria - e, mi sembra, anche abbastanza volgare - il decreto delle donne. È stato esaminato e discusso dalla Camera dei deputati nel giro di un paio d'ore. Io, invece, ritengo che tutte le volte che un decreto-legge interviene in materia elettorale sia un fatto molto grave. Dal punto di vista normativo e costituzionale, per i tempi, il buonsenso e gli effetti che produce credo si possa parlare di un vero e proprio obbrobrio. Un obbrobrio per i suoi contenuti.

si parla del mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché della legge 15 febbraio 2016, n. 20. Ebbene, peccato che nella legge a cui si fa riferimento non si parla di elezione dei membri della Giunta, che fra l'altro non vengono eletti da nessuno. Ci si è dimenticati la parola «incompatibilità»; ma in un testo di legge che riprende una normativa sarebbe molto discusso e discutibile il fatto che si usi un riferimento sbagliato nei contenuti. Ciascuna delle Camere ha un proprio Regolamento che, nella gerarchia delle fonti, può essere considerato quasi paracostituzionale. A livello dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, sul funzionamento del Governo l'equivalente è la legge n. 400 del 1988, che specificamente dice che non si può usare la decretazione d'urgenza nelle materie indicate al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione,

È vero che in passato c'è stato qualche pericoloso precedente, ma solitamente lo si faceva quando c'era l'accordo di tutte le forze politiche, e qui nessuno è stato consultato, oppure si è intervenuti sul procedimento E se qualcuno interviene sulla composizione delle liste - e, di più, quando si esprime la preferenza - vuol dire che si incide su quella parte che trasforma il voto in eletto; quindi è completamente al di fuori di un discorso costituzionale. Prima ho parlato di riferimenti temporali. La base di questo provvedimento è l'articolo 120 della Costituzione, ovvero laddove vengano messi a rischio l'unità giuridica del Paese oppure addirittura i livelli essenziali, i cosiddetti LEA - che la doppia preferenza possa rientrare nei LEA mi appare discutibile! - si interviene con il potere sostitutivo. La riforma che contiene l'articolo 120 è datata 2001, cioè diciannove anni fa. Quella che ha modificato l'articolo 51 è del 2003. La legge citata citata erroneamente, che contiene i princìpi fondamentali a cui si deve far riferimento nelle elezioni regionali, è del 2004, con l'aggiornamento del 2016 rispetto alla promozione della parità di accesso alle cariche elettive. Sono

23 luglio 2020 scoprendo l'urgenza nel bel mezzo degli esiti della pandemia, con i problemi che abbiamo davanti (sciopero generale per il mancato blocco dei licenziamenti,

Questo decreto-legge secondo me non solo non si poteva fare, ma è un pericolo rispetto alla regolarità delle elezioni, perché se si interviene sulla modalità di espressione del voto per tutte le altre Regioni, anche a livello di quote di lista, se sto raccogliendo le firme e ho centottanta giorni di tempo per poterle raccogliere, devo andare a modificare una lista per cui stavo raccogliendo già le firme? Quindi, se qualcuno non presenta la lista perché non ha raccolto le firme, può chiedere l'invalidazione delle elezioni perché non è stato messo nelle condizioni di avere i centottanta giorni di tempo per raccogliere le firme? A me sembra un pericolo eccessivo

Hanno votato in Regione Piemonte? Sì. La Regione Piemonte ha mai fatto una legge elettorale con la doppia preferenza? Mai; usa la legge statale. Pertanto, laddove è lo Stato che non mette la doppia preferenza

che sia un bello *spot* propagandistico, poi *cui prodest* non so: se è fatto per riuscire a portare anche il MoVimento 5 Stelle a sostegno di Emiliano, per far ritirare la candidatura di Scalfarotto o per dare un bel calcio negli stinchi all'autonomia delle Regioni. Ministro Boccia, non si può dire di voler sostenere l'autonomia differenziata e poi con un decreto-leggere togliere quel poco di autonomia che c'era in capo alle Regioni. Qualcuno dice che questo è fatto per favorire la parità di accesso. Ve lo dice un umile e modesto conoscitore della materia elettorale:

la doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile, perché normalmente il maschio è maggiormente infedele della femmina,

Presidente, concludo con un appello e poi mi taccio. Se si aumenta la platea dell'elettorato passivo, frammentando l'espressione delle preferenze, si riduce la possibilità che la donna venga eletta. Le donne si mettano in lista, come abbiamo fatto noi

Presidente, esprimo un ringraziamento e un senso di sorpresa. Il ringraziamento è per come si sono svolti i lavori nella Commissione che ho l'onore di presiedere, dato che ci troviamo di fronte ad una legge che mira ad affermare un'importantissima questione di principio. Nella Commissione non ci sono stati, da parte di alcuna componente delle opposizioni, una contrarietà, un impedimento, qualsiasi iniziativa che costituisse un rallentamento dei nostri lavori e questo ci ha permesso di essere in Aula in tempo utile per prendere questa importante decisione. Non ci sono stati interventi in discussione generale, non ci sono stati emendamenti, non ci sono state da parte delle opposizioni dichiarazioni di voto quando si è trattato di dare al relatore a riferire positivamente in Aula sull'atto stesso. Come Presidente della Commissione, quindi, non posso che ringraziare per lo spirito costruttivo che si è dimostrato. Comprenderete, quindi, con quanta sorpresa ho ricevuto pochi minuti fa la richiesta da parte del mio Gruppo di intervenire su una pregiudiziale di costituzionalità. Diciamo che si è inserito un elemento innovativo nella procedura parlamentare: tutto mi sarei aspettato tranne che una pregiudiziale di costituzionalità, dopo che le cose erano andate in quel modo. Ma tant'è. Al senatore Calderoli, che ha illustrato le ragioni che lo inducono a ritenere incostituzionale questo provvedimento, vorrei dire che tutta la sua dottrina - che è vasta, glielo riconosciamo tutti - andrebbe messa al servizio di battaglie più nobili e più utili. Questa non mi sembra una battaglia né nobile né utile mi è sembrato estremamente pretestuoso, a parte il finale dietrologico che confesso di non avere assolutamente capito. Il punto è eminentemente politico: siamo di fronte ad un principio, quello di favorire la parità di accesso alle cariche elettive per le donne, che è fissato in maniera inequivocabile non nel solo articolo 120 della Costituzione, ma nell'articolo 117, al comma 7, e nell'articolo 51. 51. Credo che non si possa scherzare quando si è di fronte ad un caso come quello rappresentato dalla vicenda della Puglia e credo che il Governo avrebbe sbagliato a non creare le condizioni per esercitare i poteri che gli attribuisce l'articolo 120 della e penso che l'abbia fatto rispettando i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà che in quell'articolo sono citati. Come ha detto la senatrice Valente nella sua relazione, il Governo non ha agito dalla sera alla mattina, ha invitato ad adeguarsi, ha diffidato e quando non aveva altri strumenti ha usato quello dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Ma dirò di più: non solo non c'è alcun elemento, nel provvedimento, che possa autorizzare un'accusa di non conformità alla Costituzione (semmai avremmo tradito i principi e i valori della Costituzione non muovendoci), ma dobbiamo dire che questo non basta e che sono necessari per favorire la parità di accesso alle cariche elettive anche altri provvedimenti. Vedo con favore quello che hanno varato i colleghi della Camera per intervenire anche sulla questione della inammissibilità delle liste che non rispettano l'equilibrio tra i generi e per intervenire anche nelle altre Regioni - perché la Puglia non è la sola - dove la doppia preferenza

per favorire la presenza delle donne in tutti gli enti che sono soggetti a nomine pubbliche. Mi auguro, dato che è stato firmato da tutti i Gruppi parlamentari, che su questo provvedimento si possano creare le condizioni per porlo su una corsia veloce e per avere un'approvazione unanime.

tutti sono pronti a sostenerla a parole, tutti si riempiono la bocca della necessità di raggiungere la parità di genere, vanno nei *talk e si fa un gran parlare, ma poi al momento dei fatti, al momento di dimostrare il vero sostegno, la convinzione sulla necessità di raggiungere la parità di genere, si dice qualcosa del tipo: care le mie donne, scusate tanto ma questo non si può fare, questo costa troppo; qui c'è già un uomo che reclama legittimamente il suo posto, quindi scusate tanto, anche per questa volta la parità di genere la conquisterete la prossima volta. *(Applausi).* È successo proprio qui anche in quest'Aula, esattamente con il medesimo copione, e stava per succedere nel consiglio regionale della Puglia. Ebbene, è dovuto intervenire il Presidente del Consiglio, esercitando i suoi poteri sostitutivi, per far valere ciò che alle donne è dovuto: il loro, il nostro posto nelle istituzioni, il nostro posto come rappresentanti e portavoce dei cittadini. Ricordiamo che nella prima legislatura della storia della Repubblica le donne elette, noi donne eravamo 49, il 5 per cento del totale; nel 2018, in questa legislatura, abbiamo raggiunto il *record* di rappresentatività perché siamo una su tre. Bene, ottimo, ottimo, ma non basta ancora e per raggiungere questo risultato ci sono voluti settant'anni. Si calcola che per raggiungere la piena parità nella rappresentatività delle cariche elettive ci vorranno altri questo episodio nel Consiglio regionale della Puglia proprio non ci voleva, perché rischia veramente di farci fare un ulteriore passo indietro, se pensiamo che per raggiungere la parità economica,

quadro, in cui i dati ancora dimostrano che il lavoro di cura pesa per il 75 per cento sulle spalle delle donne e in cui il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi in Europa e cala ulteriormente e drammaticamente dopo una gravidanza, una gravidanza, alcune forze politiche al Consiglio regionale pugliese hanno avuto il coraggio di cercare di seppellire le donne, i loro diritti e i nostri diritti sotto una vergognosa montagna

e di garantire che tutto sarebbe andato avanti come prima. Nessuno ha bisogno delle quote rosa; infatti non esistono le quote rosa, esistono le quote di genere, a tutela di entrambi i generi. Questa volta è andata bene. Questa volta è successo qualcosa che non era mai successo prima e questo vile attacco ai diritti delle donne e alla stessa democrazia è stato sventato dal Presidente del Consiglio. Ma non sempre ci sarà un Presidente del Consiglio così in futuro. L'unico antidoto affinché ciò non succeda più è allora che noi donne - lo so che è faticoso, lo so che costa sacrificio sacrificio - partecipiamo di più alla vita politica, partecipiamo attivamente; diventerà così sempre più facile nel corso del tempo e non rischieremo mai più di essere cancellate dalle procedure.

quella di oggi è una giornata importante, perché la politica si assume con convinzione l'impegno di affermare la forza di un diritto inviolabile, sancito dalla Costituzione e dalla legge della Repubblica: la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive. Questo provvedimento si carica del significato profondo con cui i Costituenti hanno inteso dettare la Legge fondamentale dello Stato: la volontà di non fermarsi all'enunciazione dei diritti e dei princìpi su cui poggia la nostra democrazia, ma di andare oltre, per ribadire l'importanza capitale della loro difesa e realizzazione, mettendo nuovamente in piedi e rinsaldando la logica della responsabilità, per riaffermare così la qualità della democrazia, l'immagine e la credibilità del nostro Paese. Oggi l'azione di questo Parlamento assolve pienamente a quel dovere e, grazie a questo intervento, si restituisce anche alle elettrici e agli elettori pugliesi la facoltà di liberarsi e soprattutto di esprimersi liberamente e pienamente. una questione che il Governo nazionale, il Governo della Regione Puglia e il suo Presidente e il Partito Democratico hanno sempre ritenuto centrale, e lo dico da pugliese. Si tratta di un essenziale passo avanti per i diritti delle donne, che chiama in causa una visione del mondo, la prospettiva della modernità, dei diritti umani, che sono diritti politici, civili e sociali, che intendiamo realizzare anche attraverso decisioni forti e ampiamente condivise, come la proposta di legge presentata a prima firma dalla senatrice Pinotti e sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari, insieme. È anche questo, dunque, un passaggio importante che merita rispetto e condivisione politica, avendo al centro una battaglia di civiltà, e che necessita di una convergenza che vada oltre l'appartenenza partitica e si realizzi attraverso scelte nette e, dunque, identificabili. È un passo avanti, ma non è sufficiente per dire vinta questa battaglia di civiltà. La parità di genere, il tema della giusta rappresentanza delle donne nelle assemblee e nei ruoli di guida è ancora una questione viva e pulsante su cui c'è ancora tanto da lottare e non può essere aggirata attraverso le strategie di chi, di volta in volta, tradisce esattamente la volontà di non procedere: un atteggiamento deleterio per l'intera comunità che rende anche livida la funzione e gli impegni stessi che la politica deve assumere su di sé. una lotta che, purtroppo, ancora oggi viene a volte svilita, arrivando anche a manifestarsi in una vera e propria rimozione di genere, come ha acutamente detto il ministro Provenzano; una lotta che apre un varco nel muro di indifferenza contro cui spesso si infrangono le ragioni delle donne. Questa è una tra le questioni più salienti e urgenti da affrontare nel nostro tempo. È questo un punto politico di fondo, una necessità morale che riconosca il valore del confronto con le competenze, con le sensibilità diverse e con i linguaggi nuovi che l'universo femminile quotidianamente mette in campo. È questa una priorità culturale che necessita di determinazione e di coraggio. Eppure, anche nel tagliare questi traguardi di civiltà, si incontrano spesso resistenze ostinate e fuori dal tempo. Riacquistare dignità in tema di rappresentanza istituzionale è fondamentale; mai come in questa fase critica è essenziale per continuare a mettere in campo risposte di sostanza per tutte quelle donne che oggi vivono dimensioni di difficoltà. Tempi e spazi nuovi sono necessari, rivisitati attraverso un cambio effettivo di paradigma. In una realtà in cui mai come ora le relazioni umane si intersecano in una rete caratterizzata dalla fluidità e dalla debolezza dei legami intersoggettivi, ancora più importante e urgente è risolvere queste contraddizioni e colmare questi vuoti. Un passaggio, quello che si compie oggi, necessario e urgente, che incrocia ed interpreta gli snodi essenziali delle moderne democrazie; un passaggio che sia ancora alla solidità dei princìpi costituzionali ispirati ad una logica di costruzione sociale. Attraverso un impegno serio, certo e maturo, i diritti delle donne possono e devono acquisire quella pienezza ed inalienabilità in grado di ergere il rispetto della dignità umana al di sopra di ogni contingenza. Sono questi indispensabili salti di civiltà, necessari a non farci piombare nella notte della politica e, dunque, nella notte della Repubblica.

Innanzitutto, l'avvio della discussione ci ha sorpreso, perché non avevamo previsto neanche noi come Gruppo la questione pregiudiziale e difatti non abbiamo partecipato sostanzialmente al voto.

noi vorremmo che presto, in un futuro non troppo lontano, norme che facilitino l'ingresso delle donne in politica non debbano più avere ragione di esistere, per il semplice fatto che con la raggiunta parità dei generi non avrebbe

di valere per quello che dimostra, in politica come in tutte le altre professioni. Ma oggi - lo abbiamo sempre sostenuto - una norma del genere è comprensibile. Peraltro, la mia formazione politica credo non abbia bisogno di dare dimostrazioni. Siamo l'unico partito che ha come *leader* una donna e siamo un Gruppo che ha come vice presidente del Gruppo una donna. Potrei citare esempi anche antichi: quando ero neo deputato e coordinatore regionale della Lombardia, il partito indicò una donna come vice presidente della Regione; era la massima carica che in quel momento aveva la destra politica italiana in Lombardia e addirittura in Italia. Intervengo perché non mi è piaciuto l'intervento della senatrice Maiorino. La senatrice Maiorino è ignorante, nel senso del verbo «ignorare», perché non conosce la situazione in Puglia. Io sono stato in Puglia e mi sono documentato molto bene, senatrice. molto bene, senatrice. Tutti e tre i Gruppi di centrodestra hanno detto al Presidente della Regione Puglia di essere totalmente a disposizione

Ciò che mi interessa è la genesi della vicenda in Puglia, dove non ci sono parti politiche a sostegno e parti politiche non a sostegno, al contrario - si piega un problema come questo all'opportunismo del momento e questo è male e un danno per gli uomini, le donne, la politica e la parità decreto-legge si sarebbe potuto benissimo evitare se il Governo di centrosinistra della Puglia non avesse cercato di utilizzare la questione della parità di genere per altri fini e insistendo. Ripeto, non ci sarebbe stato bisogno di forzare le norme con un decreto-legge in materia elettorale che non ha precedenti, ma che noi accettiamo come conseguenza dell'errore del centrosinistra pugliese che ha costretto il Governo a questa eccezionale

confermando la speranza di un tempo vicino in cui non sarà più necessario considerare le donne un genere che ha bisogno di un supporto.

il momento in cui non ci sarà bisogno di difendere la presenza delle donne non solo in Parlamento, ma in tutti gli organismi (penso al mondo universitario e a quelli della ricerca e dell'impresa), perché la qualità specifica del contributo femminile si impone all'attenzione per i frutti e per ciò che è in grado oggettivamente di dare. Io stessa, per l'età, per i capelli bianchi e per tutto ciò che questo significa, non ho mai goduto del fattore agevolante della quota rosa. Tutto quanto è stato frutto di un lavoro, di una fatica, di uno sforzo di convinzione e di coinvolgimento. Ma, proprio perché in questo momento, per la mia storia personale e per la storia delle persone che mi sono accanto,

grazie a tutti che supplisce a ciò che percepisco come un pregiudizio, e quindi anche come un'ingiustizia, attraverso un riconoscimento a priori del merito, ed è quello che fissa in qualche modo le quote. Certamente mi ha colpito molto l'*iter* del provvedimento al nostro esame. Francamente tra la folla di decreti da cui siamo stati schiacciati e soffocati dall'inizio del *lockdown* ad oggi, non si sentiva il bisogno dell'ennesimo decreto. Mi ha colpito anche molto la velocità assoluta con cui si è stabilita una sintonia tra il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni e il voto. Mi piacerebbe che - come accaduto con il ponte di Genova

ma allora che lo si faccia, perché l'elemento veramente dissonante in questo momento è che lo si sia fatto solo per il provvedimento al nostro esame. Il Presidente del Consiglio non dica che non si può fare. Dica piuttosto quando e come e se si vuole fare, perché i problemi urgenti di questo Paese sono tanti. Ne cito uno che ci sta travolgendo, che è quello che riguarda la scuola, ambito in cui la confusione sembra aumentare con una sorta di entropia negativa. Ogni volta che si interviene, la confusione aumenta, senza che questo contribuisca in alcun modo a dare rassicurazione alle famiglie e ai genitori. Il Governo è in grado di prendere decisioni e allora identifichi bene tutti i suoi obiettivi. Non che il provvedimento al nostro esame non sia un obiettivo in questo momento, ma sicuramente non è l'unico. Ciò che lo rende fazioso, in qualche modo, è il fatto che costituisca un'eccezione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è una giornata storica per i diritti politici, in particolare per i diritti di noi donne pugliesi. Il Governo e il Presidente Conte, mostrando particolare sensibilità alla problematica, dovuti intervenire con apposito decreto-legge per adeguare la legislazione della Regione Puglia ad una norma approvata in Parlamento nel 2016 che, appunto, prevede il vincolo della doppia preferenza. Solo agli elettori pugliesi era stata negata la garanzia di poter scegliere tra candidati di diverso sesso, così come avviene in tutte le Regioni d'Italia, in occasione della competizione elettorale imminente. devo constatare, da pugliese, come il Consiglio regionale non abbia posto tempestivamente rimedio a questo *vulnus*, riducendosi all'ultima seduta utile, dopo la diffida del Governo, per approvare questa normativa prima dello scioglimento dello stesso Consiglio regionale. In realtà, per giochi di potere di uomini tra destra e sinistra, tra emendamenti vari e mancanza di numero legale, si era si era realizzato un nulla di fatto. È stata la prima volta che un Consiglio dei ministri abbia dovuto sopperire a tale inadempimento, esercitando i poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione per ripristinare uno stato di diritto che mira ad eliminare qualsiasi disparità di genere. Con forza posso affermare come solo il MoVimento 5 Stelle abbia lottato fino alla fine per portare questo risultato, tenendo presente che, già a livello regionale, su otto consiglieri tre sono donne. *(Applausi)*. Da un'analisi della Corte costituzionale, compito della Repubblica è la rimozione degli ostacoli socio-economici, sulla base di interventi pubblici che mirano, da un lato, a sostenere le categorie svantaggiate di cittadini e, dall'altro, ad estendere a tutti, uomini e donne, la partecipazione alla vita politica, economica e sociale. Citando le parole di Bobbio, l'uguaglianza intesa come uguagliamento dei diversi è un ideale permanente e perenne degli uomini viventi in società. Ogni superamento di questa o quella discriminazione viene interpretata come una tappa del progresso civile. Orgogliosamente, oggi posso affermare senza remore che, con il decreto in esame, stiamo realizzando in pieno un'altra tappa per il progresso civile del nostro Paese. Un rinnovamento della politica e della società si realizza con il contributo congiunto e con una partecipazione equilibrata di donne e uomini. La partecipazione ugualitaria delle donne, a tutti i livelli delle strutture decisionali, in campo economico, sociale e culturale è necessaria per garantire le esigenze di entrambi i sessi nelle politiche, nei programmi e nelle azioni. La giornata del 28 luglio per la Puglia rappresenta un momento buio, dove all'improvviso sembrano vanificarsi le lunghe battaglie sostenute dalle donne partigiane che riuscirono ad ottenere l'incarico pubblico per una donna. una donna. La presenza femminile nelle istituzioni rappresenta il raggiungimento di una democrazia compiuta e garantisce la rottura di vecchi sistemi di potere. Io sono un dirigente penitenziario, un direttore di carcere, e posso attestare che la presenza delle donne, in questo ambiente prevalentemente maschile, garantisce quella sensibilità appartenente solo alla sfera femminile. La democrazia paritaria è ciò a cui il nostro sistema deve tendere e rappresenta una questione di civiltà giuridica. Proprio per questo, la democrazia paritaria non è né una concessione né un regalo.

Come senatrice del MoVimento 5 Stelle mi pregio di far parte di un Gruppo che detiene il più alto numero di presenze femminile tra le sue file: una dimostrazione pratica di come la politica può farsi attraverso la parità dei diritti tra uomo e donna e possa aumentare quei livelli, ancora troppo bassi, della presenza delle donne nelle cariche istituzionali a tutti i livelli.

il Consiglio regionale della Puglia è composto da 50 consiglieri regionali - le donne sono cinque su 50 la Giunta regionale della Puglia, composta da nove assessori più il presidente, vede la presenza di una sola donna. La relatrice, nel suo intervento, prima ricordava che, a livello nazionale, la media della presenza femminile negli organismi

è che non c'è stata capacità, da parte degli organismi di quella Regione, di arrivare in maniera autonoma a potersi dare delle regole e delle norme che potessero garantire la parità di genere nell'espressione del voto da parte degli elettori pugliesi.

possibilità di stoppare l'*iter* del provvedimento, credo proprio venga meno. Del resto, l'articolo 120 della nostra Costituzione parla in maniera chiara della possibilità data al Governo di intervenire, in maniera sussidiaria sussidiaria e rispettosa del principio di leale collaborazione, al posto di una Regione, per garantire la tutela dell'unità giuridica. Posto che, prima dell'emanazione del decreto in esame, il Governo ha tentato a più riprese di collaborare lealmente con la Regione Puglia, per arrivare alla definizione di questo principio e posto che ha lasciato tutto lo spazio e il tempo necessari affinché il Consiglio regionale potesse adempiere all'obbligo in questione, esercitando pienamente la propria funzione,

anche nella Regione Puglia, come nel resto del Paese, le donne abbiano la possibilità di accedere in maniera paritaria, come gli uomini, alle cariche elettive, per un principio che potremmo definire "paradosso delle priorità". È, cioè, ormai appurato e verificato che persone diverse e di genere diverso

la specificità di genere, la storia che ciascuno ha alle spalle e le sensibilità che la natura attribuisce a ciascuno di noi aiutano ad arrivare a determinazioni più precise, più complete più rispettose delle esigenze di molti, anche di chi magari, a volte, non viene adeguatamente rispettato.

È una cosa che mi ha colpito, è molto bella e credo che molti di noi facciano politica, interpretino il proprio ruolo e si sforzino di agire nel loro servizio servizio alla Nazione, al Comune o alla Regione, cercando di farlo "insieme", per quanto possibile, anche rispetto alle differenze politiche che pure ci sono. Ecco, forse a volte quest'insieme andrebbe declinato proprio a partire dai differenti generi e non soltanto insieme alle diverse forze politiche o alle varie anime che abitano una stessa comunità politica. Riuscire davvero nello sforzo d'includere uomini e donne nei processi; farlo farlo - certo - partendo dalle norme, ma poi permettendo ai cittadini di esprimere liberamente una tale scelta; e, quando si eleggono un sindaco o un presidente di Regione, che le norme li aiutino a garantire che quest'insieme si traduca in una presenza equilibrata

in linea generale non amo gli interventi normativi che tendono a stravolgere e cercano di plasmarla, a volte fino a deformarla. In questo senso, le quote rosa tecnicamente regole per la parità di genere, rosa o azzurro che sia, ma sappiamo tutti che di quote rosa si tratta - possono essere accettabili se si configurano come aggiustamenti temperati e soprattutto circoscritti nel tempo; insomma, se si tratta di incoraggiare fenomeni che possono portare a un miglioramento della società. Se invece s'intende la legislazione in materia come uno strumento di ortopedia sociale per l'introduzione di un gesso permanente, il discorso cambia e, in questo caso, sarei decisamente contrario. L'intervento sulla legislazione elettorale della Puglia a me pare, in questo senso, *borderline*: non serve infatti ad assicurare spazi nelle liste, già erano garantiti, ma in qualche modo a incoraggiare l'espressione di un voto, seguendo una direzione esistente ormai un po' dappertutto. Non è tuttavia di questo che voglio in

sa di doversi regolare tenendo conto che nelle liste ci sono uomini e donne; per arrivare infine anche all'esercizio eventuale del mandato nelle Assemblee rappresentative, il cui equilibrio di genere leggi come queste evidentemente intendono favorire. In queste stesse ore, però, la vostra maggioranza medesima sta sostenendo nell'altro ramo del Parlamento una legge che, nel combinato disposto tra il suo articolato e i testi illustrativi, in qualche modo nega l'oggettività dell'identità sessuale e fa assurgere il suo esatto opposto, ossia un'identità di genere fluida e sganciata dal dato biologico, addirittura a diritto inviolabile dell'uomo, protetto dall'articolo 2 della Costituzione. Questo è ciò che si evince dalla relazione illustrativa. Le due iniziative a me paiono in evidente contrasto. Lo dico per paradosso, ma neanche poi troppo: che succederebbe se una persona computata come donna nella compilazione delle liste il giorno dopo si professasse uomo? Prevarrebbe la tutela della parità di genere, perseguita da questo decreto-legge, o il diritto all'identità di genere, sancito dalla legge in discussione alla Camera? C'è evidentemente un problema, il quale - sia chiaro - non ha nulla a che fare con quella che, nel senso comune, viene definita omofobia. Una cosa, infatti, è la libertà di scelta nelle preferenze sessuali che, per quel che mi riguarda, è fuori discussione e della quale ciascuno risponde ai propri dettami. Altro è svincolare l'identità sessuale - che, per inciso, è presupposto stesso perché l'opzione omosessuale abbia un significato anche dal punto di vista semantico: se nego l'identità, evidentemente nego anche l'omosessualità - da un dato di oggettività. tutto ciò pone in evidenza un conflitto tra scelta sessuale e identità sessuale. E non è un caso che tale conflitto sia deflagrato in questi giorni all'interno dello stesso mondo LGBT e tra una parte di esso e il mondo femminista, che dopo anni di battaglie per la parità come quella che ha portato al decreto che stiamo discutendo oggi - vedono gli spazi conquistati messi in dubbio da un'ideologia che contesta il presupposto stesso (cioè, l'identità sessuale) del loro riconoscimento. Con risvolti Con risvolti anche assai pratici: è ad esempio notizia di queste ore che in altre parti del mondo vi sia una sollevazione delle atlete donne contro le *trans*-atlete, ovvero contro la possibilità che atleti uomini

Colleghi della maggioranza, vi do un consiglio: leggetevi gli scritti della Rowling, la mamma di Harry Potter, e le reazioni che essi hanno suscitato. Colleghi, dovete compiere una scelta: sostenere oggi l'identità sessuale o annegarla domani nell'acido del *genderfluid.* In caso contrario, incorrerete in un'insanabile contraddizione che si farà, per forza di cose, contraddizione normativa. Non è un problema da poco. E, forse, è un problema di cui vale la pena che il Parlamento discuta. *(Applausi).* PRESIDENTE.

la legge regionale che richiamasse i principi di parità di genere. Non è riuscito: lo aveva promesso in tutta la legislatura come punto fondamentale del programma amministrativo e politico della Giunta di centrosinistra. Non è riuscito nella sua consiliatura

Molte volte si predica bene, ma si razzola male nei fatti: il centrosinistra predica bene sui diritti civili e sulla parità di genere, ma nei fatti non è in grado assolutamente di far approvare alle proprie maggioranze una legge elettorale, come in questo caso è accaduto in Puglia.

120 della Costituzione, che consente al Governo di sostituirsi alle Regioni e agli enti locali, viene utilizzato solo in determinati casi, e sappiamo tutti quali sono: il mancato rispetto di norme e trattati internazionali, il pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica. Sono tre casi gravissimi citati nella nostra Costituzione e, quindi, nello specifico, possiamo dire che la Regione Puglia non ha rispettato il terzo punto, ovvero i i princìpi della tutela dell'unità giuridica; pertanto, una responsabilità, come dicevo, politica, ascrivibile soltanto al Governatore pugliese.

e oggi ricorriamo a uno strumento molto insolito che può creare veramente difficoltà nel nostro Paese e soprattutto nei rapporti tra Stato e Regioni. Signor Presidente, senatrici e senatori, quest'oggi siamo chiamati a discutere ed esprimerci sul decreto-legge in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali a Statuto ordinario. L'eccezionalità, direi lo stile di questo Governo si manifesta anche in questa occasione intervenendo di imperio nel delicato ambito dei regolamenti regionali e in ragione dell'attenzione a un principio basilare di cui non dovremmo stare qui a parlare, cioè quello di rendere effettiva e tangibile la parità di genere anche nella Regione Puglia, in questo estremo lembo di terra che è terra d'Europa. Ciò rende urgente e improrogabile il decreto-legge in esame, che - ricordiamoci - giunge come atto finale alle numerose richieste da parte dello Stato centrale, espresse a mo' di raccomandazione. Non è tanto l'approssimarsi dell'appuntamento elettorale - certo, anche quello, perché non risolvendo rischiamo di rimandarlo per altri cinque anni - quanto il fatto di dare maggiore impulso alla ricucitura del *gap* di genere intollerabile in un Paese civile del XXI secolo come l'Italia. attuale è il tempo delle decisioni forti, e il nostro attuale Governo ha tutta l'autorevolezza e la stima per poterlo esprimere con questo ulteriore atto, in conformità dello spirito costituzionale, come formulato nell'articolo 3 della nostra Costituzione, e che vollero fortemente le nostre madri Costituenti, e così pure i padri, tanto da averlo collocato tra i primissimi articoli del testo. testo. Quello che faremo oggi altro non sarà se non l'adempimento di una promessa fatta più di mezzo secolo fa, rimasta disattesa per troppo tempo. Mi auguro che non resti un caso isolato, un *unicum*, ma invece sia il preludio di una nuova stagione di cambiamenti anche per le altre Regioni, che ancora ricalcitrano ad ammettere il nuovo stato delle cose. Ritorniamo alla terra di Puglia, terra magica che ha espresso il tarantismo, un fenomeno complesso antropologico con cui soprattutto le donne hanno imparato nei secoli a esprimere il loro malessere esistenziale e con cui hanno preteso attenzione, come mirabilmente ha spiegato lo studioso Ernesto De Martino nel suo saggio del 1959 «La terra del rimorso». Oggi le donne hanno finalmente canali istituzionali con cui potersi esprimere, e sicuramente quello di garantire la loro giusta presenza nelle istituzioni è un segnale forte per giungere alla parità di genere, soprattutto per le donne pugliesi in quanto, oltre a essere numericamente di più (il 51 per cento), hanno anche un livello di scolarizzazione più elevato. Ecco, dunque, che il tema della rappresentanza viene a legarsi a quello della presenza paritaria femminile. Questa è la democrazia. È uno scatto di orgoglio femminile che si allega a quello di uomini che sono già maturi e pronti per il cambiamento; se volete, un atto di protesta proprio come è stata a lungo la tarantella, ma in forma più composta. *(Applausi).*

coraggioso, il quadro normativo richiamato (gli articoli 120 e 122 della Costituzione e l'attuazione della legge n. 165 del 2004, così come modificata nel 2016) consente questo intervento. Mi permetto adesso di soffermarmi brevemente sul tema tema oggetto del provvedimento, anche in relazione ad alcuni interventi che mi hanno sollecitato.

la stigmatizzazione di un comportamento che rischia di penalizzare le donne e quindi l'impegno ad adoperarsi affinché, insieme ad una legge che di per sé è necessaria ma mai sufficiente, si cambino anche comportamenti, pratiche e culture che rendono oggi difficile l'accesso delle donne alla vita politica e istituzionale; un accesso - lo ricordo - molto difficile in generale e molto complicato

c'è una norma antidiscriminatoria, che è una cosa ben diversa dalla quota, che è un orientamento assolutamente accreditato in sede internazionale, così come in sede nazionale. Noi ci stiamo adoperando ad adottare una norma antidiscriminatoria, com'è stato richiamato in più interventi. Nessuno dei due generi deve essere sottorappresentato nelle liste e, dall'altro lato, diamo una possibilità in più all'elettore di esprimere la preferenza. Ampliamo le possibilità dell'elettore, non le restringiamo. Del resto, se annulliamo, annulliamo solo la seconda preferenza; quindi non restringiamo il campo, ragion per cui la Corte costituzionale si è pronunciata a favore della legge elettorale della Campania e di tutte le altre che si sono susseguite. Mi permetto infine di dire che il provvedimento che oggi stiamo per assumere interviene direttamente sulla qualità della democrazia e non è una concessione che facciamo alle donne. È una battaglia che conduciamo per la qualità delle nostre istituzioni democratiche, intanto perché siano più più democratiche di quanto non lo siano state fino a questo momento e perché la partecipazione delle donne, anche grazie alla doppia preferenza, ha cambiato notevolmente in nostro Paese. Questo Parlamento ha cambiato volto grazie alla possibilità, attraverso lo strumento delle primarie, di arrivare con la doppia preferenza, e anche le Regioni hanno cambiato volto. Cambia anche la qualità del prodotto dei luoghi della democrazia in questo Paese, quando a partecipare a pieno titolo sono le donne e gli uomini.

non è di rito, ma è sentito da parte di tutto il Governo, perché in pochissimi giorni il Parlamento si appresta a convertire in legge un decreto che il Governo stesso - senatore Quagliariello - non avrebbe voluto emanare. L'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 è stata spesso richiamata e richiesta, in questi mesi drammatici, e il Governo ha sempre tentato, fino all'ultimo, la mediazione con le Regioni. Lo abbiamo fatto su tanti temi di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione, dalla sanità ai trasporti, nei momenti più difficili e drammatici che riguardavano anche l'ordine pubblico, alla fine sempre di comune accordo con le Regioni. E, che il presidente Mattarella sempre ci ricorda della leale collaborazione, abbiamo trovato una soluzione. Questa volta non è stato possibile - voglio dirlo soprattutto ai colleghi intervenuti dai banchi dell'opposizione

hanno non solo accolto la mia prima lettera, che a nome del Governo invitava i Consigli regionali restanti ad adeguarsi, ma di fatto hanno anche chiesto indirettamente che l'intervento del Governo fosse conseguente se i Consigli regionali non si fossero adeguati. Voglio ricordare qui in Aula - lo ringrazio tutto - che il Consiglio regionale della Liguria, dopo la diffida, ha adeguato all'unanimità, con un dibattito alla luce del sole,

ricordare - spesso ritroviamo anche nei dibattiti parlamentari: si dicono alcune cose, e poi se ne fanno altre. E, quando si richiama - come è successo purtroppo spesso nella storia recente di quel Consiglio regionale - il voto segreto per rispondere

in quel Consiglio non c'erano le condizioni e alla fine siamo intervenuti. E lo abbiamo fatto perché era inevitabile intervenire e lo faremo anche per il Piemonte e per la Calabria. Qualcuno qui in Aula, signor la Calabria. Il senatore Calderoli, il cui saluto affettuoso ricambio, e con il quale abbiamo condiviso molti momenti in queste Aule, con la sua nota competenza ha ha ricordato che il Governo non è intervenuto nello scorso aprile, ma è cambiata la maggioranza - lo dico con grande franchezza - ed è cambiata anche la sensibilità su questi temi. Con il Presidente del Consiglio abbiamo posto un tema chiaro: o si fa, o si diffida. La Regione Liguria l'ha fatto e abbiamo ringraziato il presidente Toti e tutto il Consiglio regionale dal Governo e l'ho fatto personalmente in Conferenza Stato-Regioni. Piemonte e Calabria non lo hanno fatto e, se non lo faranno, interverremo noi con un atto sostitutivo, ma sono sicuro che Piemonte e Calabria lo faranno. La stessa presidente Santelli, che dimostra come una donna possa guidare una Regione del Sud e cambiare il corso della storia e degli eventi, prende atto che sono solo tre le donne presenti nel Consiglio regionale della Regione Calabria. I Comuni, da quando ci sono le norme sulla parità di genere, hanno più che triplicato la presenza delle donne nei Consigli comunali.

alcuni contestarono l'intervento. Grazie a quell'intervento oggi è cambiata la rappresentanza. Non c'erano donne allora? Certo che c'erano, erano all'altezza ed erano anche più brave. Oggi ci sono e guidano quei processi.

ha accettato l'intervento fatto dal Governo, ringrazio ancora i Gruppi per i contributi che ci hanno dato in discussione generale e chiedo che venga trasmesso al Senato anche il parere che l'Avvocatura generale dello Stato, su richiesta del Governo, aveva approntato, perché penso che il passaggio che l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto sull'unità giuridica e sulla parità di genere sia un grande contributo al nostro dibattito.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, dove c'è una discriminazione c'è qualcuno che ne trae un privilegio. È questa la ragione per cui le resistenze a norme come quella in esame sono sempre molto alte. In Puglia la normativa sulla doppia preferenza è stata vittima di una gigantesca ipocrisia, perché il partito contro le donne non conosce colore politico: prima la maggioranza ha calendarizzato il provvedimento l'ultimo giorno utile, lanciando così un chiaro segnale a un consiglio composto al 90 per cento poi sono arrivati 2.000 emendamenti ostruzionistici dell'opposizione che hanno creato il terreno ideale per far mancare, nel cuore della notte, il numero legale. In questo modo tutti hanno avuto la possibilità di scaricare la colpa sugli altri, ma in realtà sottobanco potevano festeggiare tutti quanti.

Gli argomenti per giustificare la contrarietà alle azioni positive sono tanti e purtroppo ci sono anche molte donne a sostenere di non essere una specie in pericolo di estinzione, che chi ha le competenze non ha bisogno di aiuto, che le azioni positive sono una umiliazione per il nostro sesso. Purtroppo non è così. Le donne hanno sulle loro spalle secoli di discriminazione e in Italia solo con la Costituzione del 1948 viene inserito per la prima volta il principio di uguaglianza tra i sessi nell'ordinamento giuridico; solo dal 1963 le donne sono state ammesse a tutte le professioni, per esempio al concorso in magistratura, e solo dal 1975, con il nuovo diritto di famiglia, sono stati sanciti uguali diritti per i coniugi; poi, nel 1956, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dello *ius corrigendi* e nel 1968 quella del trattamento differenziato dell'adulterio;

che tra l'altro è rimasto un principio teorico. Si è dovuto attendere il 1981 per cancellare dal codice penale l'attenuante per i delitti d'onore. Insomma, la parità formale è stata raggiunta solo a partire dagli anni Novanta, ma tutte le statistiche ci dicono che siamo ben lontani dalla parità sostanziale. Soprattutto nei Paesi dell'Europa meridionale c'è ancora un grande divario tra i sessi. In Italia l'occupazione femminile è tra le più basse d'Europa con una percentuale di donne che hanno un impiego di 20 punti inferiore a quelli degli uomini. Solo nel 2019, 37.000 donne hanno lasciato il loro lavoro dopo la nascita di un primo figlio. Per non dire del numero ridotto di donne che ricoprono ruoli dirigenziali dirigenziali nella pubblica amministrazione e nella giustizia, nonostante queste rappresentino più della metà della forza lavoro del settore pubblico. Covid-19, poi, ha aggravato le disuguaglianze di genere, facendo pesare sulle donne l'intera gestione familiare. Particolarmente grave è lo squilibrio della rappresentanza politica. In Parlamento noi donne siamo il 35 per cento del totale e questo è il miglior dato della storia repubblicana. Nei Comuni la presenza femminile è di circa il 30 per cento, mentre nei Consigli regionali i numeri sono di regola più bassi. Il paragone con altri Paesi europei ci dimostra che in nessuno di questi un avvicinamento alla parità si è raggiunto senza azioni positive, solo che in questi Paesi le misure sono state prese cinquant'anni fa; col risultato che, ad esempio, nei Paesi scandinavi la parità della rappresentanza politica è ormai raggiunta. Nasce così l'esigenza di prendere misure correttive di discriminazione positiva, come quella che oggi stiamo votando. A imporcelo è l'articolo 51 della Costituzione, il quale sancisce che, per garantire a tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, l'accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, la Repubblica promuove le pari opportunità tra gli uomini e le donne. Da qui una serie di interventi normativi sui sistemi elettorali, tra cui la legge n. 20 del 2016 sull'equilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli regionali, con cui si impone alle Regioni di prevedere almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso. È questa la norma a cui la Puglia non si è adeguata e, come autonomista, dispiace che lo Stato sia stato costretto ad intervenire, esercitando per la prima volta il potere sostitutivo. Ma dispiace anche che questo intervento si sia limitato solo alla doppia preferenza, senza prevedere l'esclusione per le liste che non rispettano la quota di genere. In teoria, potrebbero esserci liste di soli uomini, che verrebbero sanzionate solo con un'ammenda pecuniaria. I dati dimostrano che solo se si abbinano diverse misure si registra una crescita sostanziale delle donne elette: quindi, quota di genere sulle liste, alternanza uomo-donna nell'elenco delle candidature e doppia preferenza. Dispiace anche che nella mia Provincia autonoma, nonostante le richieste delle donne, non si sia riusciti a introdurre l'obbligo dell'alternanza di genere nel voto di preferenza. Siccome il nostro sistema elettorale prevede fino a un massimo di quattro preferenze, che tradizionalmente vengono usate, sarebbe stato un intervento molto efficace; per alcuni, forse, fin troppo. Infatti, come dicevo prima, la discriminazione crea sempre un vantaggio per qualcuno e ogni postazione occupata da una donna è una postazione tolta a un uomo. In ogni caso, come Gruppo Per le Autonomie crediamo nell'importanza delle azioni positive, ma pensiamo anche che la Puglia non abbia reso un buon servizio a coloro che credono nel valore delle autonomie locali, anche quando si tratta di Regioni a statuto ordinario. Per tutte queste ragioni, esprimeremo un voto favorevole.

della doppia preferenza di genere: abbiamo una storia che ci vede costantemente favorevoli. In tutte le Regioni abbiamo proposto e votato ogni legge elettorale che prevedesse la doppia preferenza di genere. Ricordo che anche nella mia Umbria, all'epoca, noi fummo quasi precursori e una delle proposte fu a mia prima firma e devo dire che, trasversalmente, il favore a una proposta sulla doppia preferenza di genere non era proprio così

recente tornata, come Jole Santelli in Calabria e Donatella Tesei nella mia Umbria. Quindi su questo sgombriamo il campo in ogni modo: non abbiamo bisogno di dimostrare che siamo a favore della doppia preferenza di genere come riconoscimento di una parità

cento, come stabilisce la legge, ma noi, in genere, in tutte le Regioni abbiamo elaborato liste che prevedono metà e metà. Detto ciò, il problema è la solita mistificazione dei fatti. In Puglia, colleghi, il problema non è stato istituzionale, non è stato è stato del consiglio regionale e non è stato delle forze politiche presenti in quella Regione: il problema è del PD, che oggi viene qui a farci anche la lezioncina, come al solito. È il PD che non è riuscito a far approvare una legge in Puglia che prevedesse la doppia preferenza di genere. È il presidente Emiliano che in Puglia non è riuscito a coordinarsi con la sua maggioranza, costringendola o o invitandola a votare una legge elettorale coerente con la normativa nazionale che prevede la doppia preferenza di genere. Non è un problema istituzionale, ripeto. Rispetto a questo tema, l'intervento del Governo cerca di mettere cerca di mettere una pezza rispetto alla inconsistenza e alla inesistenza di una parte della sua maggioranza. Eppure, parliamo di un partito strutturato, che viene dalla vecchia scuola; parliamo di un partito che, in teoria, dovrebbe saper trasmettere dal centro alla periferia le indicazioni di voto su temi così importanti e fondamentali.

alla forzatura di una legge nazionale che impedisce di agire sulle leggi elettorali regionali con decreto. Ci sono motivi di preoccupazione. Ma rispetto a questo, ciò che principale viene da obiettare è che il PD, che si ammanta di bandiere non sue oggi in quest'Aula, attraverso la relazione della relatrice, si ammanta di bandiere non sue - e che non riesce a trasmettere ai livelli periferici, non ci può venire a dare lezioncina, né di parità,

Le donne della Valle d'Aosta non hanno gli stessi identici diritti di parità di accesso in partenza? E come risolviamo il problema, visto che voi vi atteggiate a voler risolvere il problema della Puglia? E poi in Calabria, dove si è votato qualche mese fa, che cosa accadeva? E cosa

meno retorica e meno spocchia, perché tutti noi siamo fortemente favorevoli a mettere in campo ogni provvedimento legislativo

Ecco, rispetto a ciò, le lezioncine non le prendiamo. Quanto alle bandiere, ognuno si tenga le proprie ed evitiamo di ammantarci di bandiere che non ci appartengono.

verso l'adozione di provvedimenti che consentano alla donna di partecipare con piena parità a tutte le competizioni elettorali: con parità di partenza e non con le riserve indiane delle quote di approdo. *(Applausi)*.

nell'accesso alle cariche elettive politiche. Ne dobbiamo purtroppo ancora parlare perché, dopo settantaquattro anni di Repubblica democratica basata su noti princìpi di uguaglianza e parità sociale tra cittadini e cittadine, esiste ancora un *gap*. Molti in quest'Assemblea lo hanno detto: le donne hanno conquistato l'elettorato attivo, ma non hanno ancora pienamente conquistato quello passivo. Come ho appena sentito dire, alle donne non è ancora dato poter partecipare alle elezioni muovendo dallo stesso nastro di partenza degli uomini. Questa è la situazione.

Questa è una disuguaglianza. Le disuguaglianze persistono in Italia per motivi certamente culturali, ma anche perché molte Regioni non hanno adempiuto ai loro doveri e adottato normative rispondenti ai princìpi costituzionali di parità di accesso alle cariche elettive politiche. È evidente che l'adozione di queste norme non vuol dire garantire il risultato dell'elezione alle donne - ci mancherebbe altro - ma significa certamente promuovere la parità di accesso. «Promuovere» è un verbo dinamico e vuol dire che le Regioni devono fare, come prescritto anche dall'articolo 117 della Costituzione: è chiaro da moltissimi anni, non è che dobbiamo dirlo oggi per la prima volta.

Per quanto riguarda i sistemi di elezione proporzionali, con l'espressione delle preferenze, come nel caso della Puglia, si stabiliscono tre cose chiare, neanche particolarmente complicate: che le liste devono essere composte, almeno per il 40 per cento, dal genere meno rappresentato (non si capisce come mai non sia prevista perché mi sarei aspettata il 50 per cento, comunque siamo al 40); che si debba esprimere una doppia preferenza di genere, con libertà nell'espressione della prima preferenza, ma con la seconda preferenza che deve essere di genere diverso, pena la decadenza della seconda preferenza espressa; giustamente - le donne abbiano la stessa visibilità degli uomini nell'ambito della campagna elettorale sui mezzi di comunicazione. Purtroppo, nonostante queste previsioni siano costituzionali e siano anche molto chiare, molte Regioni non hanno adottato la normativa, oppure lo hanno fatto solo in parte.

In queste Regioni che non hanno adottato o hanno adottato parzialmente le norme sulla parità di accesso, la sottorappresentazione femminile nei Consigli regionali è evidente nei numeri.

quindi oggi è assolutamente necessario e opportuno approvare il decreto-legge in esame, per attivare il potere sostitutivo dello Stato. Quello che è interessante dirsi in quest'Aula, in modo molto chiaro, è il perché Nel corso di questi anni di impegno politico - grazie a Dio non troppi - ho capito che gli usi e le consuetudini radicate in un modello di società maschile persistono. Non me ne sono accorta solo io, tanto che ci sono scrittori e sociologi, come Aldo Bonomi, che parlano del modello sociale dell'uomo bianco di mezza età dal posto fisso, modello culturale molto radicato in Italia. persiste anche, naturalmente, perché è un modello di potere e di solito il potere si autoconserva e per autoconservarsi cosa ha fatto? Ha esercitato il potere di non scegliere di investire di non scegliere di investire risorse in servizi che avrebbero reso la nostra società, nelle Regioni e naturalmente nel complesso, realmente paritaria. Ha scelto di non investire nei nidi, di non investire nei servizi di cura, ha scelto di non investire per incentivare l'occupazione femminile, tanto che siamo fermi a meno del 50 per cento delle donne che lavorano. Queste sono scelte che pesano come macigni sul modello di Stato Italia. Purtroppo mi sono resa conto, e questo l'ho vissuto personalmente, che molte delle resistenze dipendono anche da un modello pre-culturale che definisco un po' "machista". che fu degasperiana - per fortuna lo fu, ma purtroppo non lo è più - ho sentito affermazioni irripetibili, ribadite però per ore, per creare un ostruzionismo tale da impedire l'approvazione della doppia preferenza di genere. Naturalmente, i modelli culturali prevalgono e i modelli pre-culturali soccombono e anche la Provincia autonoma di Trento ha approvato la legge sulla doppia preferenza di genere, Scusate colleghi, c'è un rumore molto fastidioso. *(Richiami del Presidente)*. Stiamo attenti perché bisogna constatare che anche le Regioni che hanno approvato la doppia preferenza di genere stanno facendo dei tentativi per retrocedere da tali conquiste con la motivazione che ci hanno provato - bontà loro - ma che le donne non si trovano. Noi lo smentiamo, allora, perché nelle liste che stiamo componendo possiamo confermare che le donne sono pienamente pronte per fare politica e naturalmente per candidarsi. che assistiamo a resistenze molto importanti dal punto di vista ambientale rispetto al tema della parità di genere e però non solo le leggi dello Stato, che ci apprestiamo anche oggi ad approvare, ma anche la Corte costituzionale ci aiuta ad andare nella direzione giusta perché ha affermato, anche recentemente con la sentenza n. 143 del 2010, che il principio della parità di accesso si applica a tutte le Regioni, anche alle autonomie speciali. Del resto, parliamo di norme costituzionali che devono essere adottate e applicate allo stesso modo su tutto il territorio dello Stato per assicurare, da un lato, naturalmente, l'esercizio pieno dei diritti politici e, dall'altro, l'unicità e unitarietà giuridica della Repubblica italiana. per usare le parole autorevoli di Martin Luther King, possiamo dire che è sempre il momento giusto per fare la cosa giusta, che non è mai troppo tardi e quindi oggi ci apprestiamo ad andare in quella direzione e a votare un provvedimento importante. Naturalmente Italia Viva vota a favore del decreto-legge n. 86 e vota a favore di ogni passo avanti verso la parità.

prima della pausa estiva, perché credo che, invece, siano state poste una serie di questioni e anche di riflessioni che meriterebbero e meritano una discussione dedicata. Provo a citarne alcune. Intanto, vorrei ricordare qui,

e soprattutto del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, in virtù del quale la Repubblica rimuove tutte le cause delle disuguaglianze, ma nel caso specifico delle delle disuguaglianze di genere tra uomo e donna noi abbiamo visto quanta sia stata la fatica, in tutta la storia repubblicana. Con questo articolo 51 si fa un ulteriore passo in avanti e voglio sottolinearlo, perché non è è cosa da poco. Eppure, noi avevamo già l'articolo 3 della Costituzione, che avrebbe già dovuto spingere tutta la legislazione repubblicana verso la garanzia dell'accesso e la rimozione delle disuguaglianze. L'articolo 51, non solo ristabilisce ancora una volta il principio che bisogna stabilire le condizioni di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive tra uomo e donna,

Fedeli. La legge n. 20 del 2016, nasce dal fatto che qui nessuno voleva comprimere la volontà di nessuno, ma spingere, quello sì, e farlo attraverso una legge nazionale in applicazione di questo principio.

non essere applicato in una parte del nostro Paese? Come riusciamo a stabilire una unità giuridica che vale per il Lazio ma anche per la Sicilia?

tema c'è e credo che questa sarà la seconda puntata che noi dovremo affrontare ed è una questione

Questo vale anche per altri principi: alcuni princìpi costituzionali non possono incontrare una barriera posta dalle dalle autonomie speciali. La questione deve essere assolutamente affrontata. Senza voler fare operazioni di alcun tipo, è un dibattito, anche costituzionale, assolutamente serio e importante. Vale anche per altri princìpi, poi un altro tema. In tutti questi anni abbiamo fatto tantissimi passi in avanti,

ci vuole, eccome! Possiamo dire che magari ci saremmo augurati fosse stato applicato anche in passato - assolutamente sì - ma che oggi ci sia è assolutamente fondamentale,

riusciamo a far compiere un ulteriore passo avanti a una lunga storia che ha questo Senato, soprattutto negli ultimi anni. Da questo punto di vista, anch'io avrei preferito non dover arrivare a quello che è stato proposto, ossia una scelta sostitutiva rispetto a quella del Consiglio regionale della Puglia, ma tant'è e ne prendo atto. Voglio ringraziare prima di tutto la senatrice Valente per la puntuale presentazione che ha fatto del provvedimento, nel merito e nella storia, che non va mai dimenticata, perché abbiamo alle spalle tantissimi passaggi.

base al quale la prima discriminazione che va superata, perché è trasversale a tutte le altre, è quella di sesso, che riguarda le donne, che sono la metà della popolazione),

importante di promozione e mi permetto di dire a mia volta in quest'Aula un concetto che mi accompagna negli anni: non stiamo parlando di quote

a questa scelta, ovviamente fortemente sostenuta dal Partito Democratico - che, peraltro, ha nel suo statuto regole e norme antidiscriminatorie; lo voglio dire a chi ci invita a riflettere sui nostri limiti - che sicuramente ci sono - ma almeno questo

seguire, secondo me, nel cambiamento. La grande lezione, infatti, che ci viene dalle Madri costituenti e da tutto il lavoro che successivamente abbiamo fatto è che, se non ci sei, non cambi le politiche. Se le donne non sono nei luoghi della decisione politica, significa che le politiche scelte non rispondono ai bisogni, ai diritti e alle necessità di metà della popolazione di questo Paese e, in questo caso, della Puglia. esserci per contare e cambiare. Questo è il grande tema che riguarda donne e uomini della Puglia e dell'Italia. Si diceva che è un tema che riguarda la qualità democratica ma anche il concetto di condividere le scelte politiche, le scelte che si fanno nell'ambito del lavoro, la genitorialità e le scelte personali. La parola «condivisione» è la grande questione che sottende a questa scelta che facciamo oggi.

all'elezione dei Consigli regionali, ma anche il tema che riguarda l'insieme delle regole di tutte le Regioni, anche a Statuto speciale. Se sono princìpi costituzionali, infatti, se sono un valore di *governance* della politica e, insieme, di condivisione, significa che ciò riguarda tutti perché è un miglioramento che serve alla Puglia e alle altre Regioni che ancora non lo hanno fatto. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, è l'occasione per parlare ancora della facilitazione dell'accesso alla politica da parte delle donne. Personalmente la mia idea non è monopolistica all'interno del mio Gruppo e Gruppo e vede le donne meritevoli di trovare dei canali di agevolazione per avvicinarle all'esercizio del diritto parlamentare, politico e manageriale negli enti pubblici. Io, però, sono contrario alle quote

se fosse stata prevista per un tempo determinato per dare la possibilità di un cambio culturale e di mentalità nel nostro Paese, ma non a una norma che reclude

esclusiva competenza regionale con un decreto-legge, cosa che non è prevista nella nostra Costituzione se non in casi eccezionali e in cui c'è stata concertazione. In questo caso, non vi è stata concertazione perché è stato un intervento suppletivo per per consentire alla Regione Puglia di vedere approvata la doppia preferenza in contrapposizione a un'incapacità di quella Regione che non è dell'ultima ora ma dura da quindici

quindi, assolutamente d'accordo nel merito; siamo contrari nel metodo. Non è un metodo giusto, non ha tenuto conto della leale collaborazione tra le istituzioni, e questo ci mette nelle condizioni di astenerci nel voto definitivo. Resta un'amarezza, quella di predicare bene e razzolare male. Concludo con una domanda: che senso ha stabilire la parità di genere nell'espressione del voto se poi non vi è una norma che garantisca la presenza delle donne nelle liste? Sappiamo, infatti, che, una volta garantita la parità di genere nel voto, le liste possono essere composte da un unico sesso e non vi è assolutamente alcuna preclusione nella presentazione delle stesse. Questo è un mistero: ci vogliamo assolvere la coscienza, ma poi non creiamo gli strumenti effettivi per realizzare realmente la partecipazione delle donne. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione del mio Gruppo su questo provvedimento.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento che stiamo esaminando mi preme sottolineare con forza e decisione che la Lega ha dimostrato a più riprese, e in maniera inequivocabile, di tenere in estrema considerazione il ruolo primario che ricoprono le donne nella politica, intesa come continua ricerca del bene comune, nel rispetto di quanto riconosciuto dalla Carta costituzionale. Lo testimoniano - solo per citare alcuni esempi - la candidatura di Lucia Borgonzoni per la guida della Regione Emilia-Romagna, quella di Donatella Tesei - attuale e ottimo governatore della Regione Umbria - o la candidatura di Susanna Ceccardi per la presidenza della Regione Toscana. *(Applausi).* È estremamente chiaro, È estremamente chiaro, quindi, che il problema del provvedimento in questione non è e non sarà mai la sua finalità, ma è lo strumento giuridico che il Governo ha scelto di utilizzare. La questione rilevante è che voi non avete alcun rispetto della Costituzione e noi, e la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, a questo non riusciamo proprio ad abituarci. Il Governo si è mosso in ritardo rispetto all'imminente scadenza elettorale che - ricordiamoci - è stata posticipata a settembre a causa dell'emergenza Covid. Infatti, l'informativa del Ministro per gli affari regionali al Consiglio dei Ministri risale al 25 giugno del 2020, mentre la diffida alla Regione Puglia è del 23 luglio 2020 e conteneva una richiesta di adeguamento della normativa elettorale regionale entro cinque giorni. Orbene, questo comporta una violazione della legge che prevede che alla Regione debba essere dato un congruo termine per adempiere. Solo in caso in cui tale termine sia disatteso è permesso al Governo di intervenire, ma sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Anche nel caso in cui l'intervento sia necessario in assoluta urgenza, il Consiglio dei Ministri dovrebbe adottare i provvedimenti necessari che devono essere comunicati alla Conferenza Stato-Regioni. L'articolo 120 della Costituzione, quindi, permette sì al Governo un intervento, ma non nei modi e soprattutto nella forma oggi utilizzata. Infatti, proprio la procedura prevista dalla legge induce a ritenere che il decreto-legge non sia lo strumento giuridico utilizzabile, in quanto vengono a mancare i presupposti previsti per la decretazione d'urgenza dell'articolo 77 della Costituzione. A ciò si deve aggiungere che l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il Governo non può provvedere con il decreto-legge nelle materie indicate dall'articolo 72 della Costituzione, tra le quali rientra la materia elettorale. Il Governo, quindi, ha ritenuto di dover intervenire con urgenza in una materia di competenza regionale, facendo venir meno il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, di fatto esercitando una clausola di supremazia che ad oggi non risulta presente nel nostro ordinamento. Tutto ciò appare come una netta testimonianza del tentativo del Governo di andare a sanare mancanze gravi del Consiglio e della Giunta regionale pugliese guidata da Michele Emiliano. È doveroso ricordare che cinque anni fa, in campagna elettorale, il governatore Emiliano promise, tra l'altro, che il primo intervento del suo Governo sarebbe stato volto a modificare la legge elettorale regionale, inserendo fin da subito la doppia preferenza di genere. Oggi, a distanza di anni, siamo qui con rammarico a constatare che quella promessa, come purtroppo altre, era solo propaganda elettorale e la fiducia che le donne avevano riposto in quella promessa è stata tradita. Quindi, non solo la rappresentanza femminile tra le fila del PD nel Consiglio regionale pugliese è scarsa, se non quasi inesistente, ma nel corso di tutta la consiliatura la maggioranza di sinistra non è riuscita a conformare conformare la legge regionale ai princìpi dell'ordinamento nazionale. *(Applausi)*. Questo sta a certificare di fatto l'inadeguatezza in questo, come in altri ambiti, del governo uscente della Regione Puglia, mentre i cittadini pugliesi meritano altro e meritano di più. Nel tentativo di sanare il fallimento del presidente Emiliano, della sua Giunta e della sua maggioranza, che per cinque anni sono rimasti colpevolmente inerti, arriva oggi un intervento statale che impone per decreto-legge alla Regione la doppia preferenza di genere nelle liste, a poco meno di due mesi dallo svolgimento delle elezioni regionali e pure a pochissimi giorni dal deposito delle candidature, attraverso un uso improprio dei dettami costituzionali, costituendo un precedente spiacevole e pericoloso del quale oggettivamente non se ne sentiva l'esigenza. I più maliziosi potrebbero vedere dietro questo intervento a gamba tesa del Governo un fine puramente propagandistico volto non perdere il voto delle donne. Il tempo ci darà risposte, ma come i saggi sempre ci insegnano «a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina». In considerazione di quanto esposto, dichiaro il voto di astensione al provvedimento del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

amore che emerge tra i banchi.

ma è anche l'anno in cui, il 10 marzo, le donne hanno votato per la prima volta. Il 1946 che ricordo qua non ha nulla a che vedere con gli anni: è il numero di emendamenti che ha presentato Fratelli d'Italia in Consiglio regionale al momento dell'approvazione della legge che modificava la legge regionale pugliese e introduceva la doppia preferenza di genere; emendamenti non ostruzionistici, a detta del capogruppo di Fratelli d'Italia Zullo. Leggo il virgolettato: «Nessun ostruzionismo; la nostra preoccupazione però è che possano essere inseriti emendamenti (...) che espongano la legge *in itinere* a rischio di incostituzionalità (...). Ritiriamo quindi tutti gli emendamenti e limitiamoci a votare il disegno di legge così come formulato in Commissione». Ma a quali emendamenti a rischio di incostituzionalità si riferivano, visto che si trattava dell'approvazione di una legge che si rifaceva alla legge n. 20 del 2016? Forse l'unico emendamento che faceva paura era quello presentato dal Movimento 5 Stelle, che introduceva la non ammissibilità delle liste con più del 60 per cento dei componenti dello stesso sesso. Poi è stato votato un emendamento di Forza Italia, chiaramente volto a bloccare la candidatura di un collaboratore di Emiliano che ha dichiarato di candidarsi con la lista a suo supporto, emendamento poi passato a scrutinio segreto anche con parte della maggioranza (credo una decina di voti).

poi, all'una e mezza di notte circa, si rientra in Aula, ma la maggioranza richiede di non proseguire, l'emendamento viene ritirato e salta magicamente il numero legale. Noi siamo qui oggi... *(Brusio)*. Presidente, non riesco a parlare... Noi siamo qui oggi a discutere e approvare un disegno di legge che non sarebbe dovuto esistere, perché è inammissibile e inconcepibile che nel 2020 siamo ancora a discutere di introdurre la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive, quasi come se fosse una concessione. Il Governo è dovuto intervenire in due tempi: prima in maniera *soft*, semplicemente facendo una diffida a intervenire alla Regione Puglia poi, quando la Regione Puglia non è intervenuta, con questo disegno di legge, richiamando agli articoli 3 e 51 della Costituzione, anzi utilizzando il dettato dell'articolo 120, che forse è la prima volta che si utilizza nella storia repubblicana. Alcuni intravvedono in questo un sopruso, una sopraffazione da parte del Parlamento nei confronti delle Regioni, io dico invece che è vergognoso che per problemi di mera esigenza politica destra e sinistra siano venute meno al dovere politico di rispettare le leggi e la Costituzione.

solo questo ed era quello che chiedeva anche il MoVimento 5 Stelle in Puglia ed è anche quello che dice l'articolo 117 della Costituzione, ovvero che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Ma che la responsabilità non sta tutta a destra, perché anche il presidente Emiliano nel 2015, appena eletto, disse che il primo provvedimento sarebbe stato quello di modificare la legge regionale ed introdurre la doppia preferenza di genere;

quindi, che in Puglia l'unico che non c'entra con questo pasticcio è il MoVimento 5 Stelle, il cui emendamento riportava alla legge n. 20 del 2016. *(Applausi)*. Tra l'altro, ricordiamo che nel 2015 il MoVimento 5 Stelle ha presentato una lista con il 46 per

Il MoVimento 5 Stelle non aveva e non ha bisogno di una legge per affermare la parità di genere, lo fa naturalmente. Chi ne ha bisogno sono gli altri Gruppi politici, che forse hanno difficoltà a candidare le donne, sicuramente in Puglia. *(Applausi)*. L'unica motivazione, quindi, è la paura degli uomini di perdere le poltrone. ci troviamo ora ad approvare questo decreto-legge che è monco di una parte importante, ovvero della inammissibilità delle liste con oltre il 60

stavano piegando le istituzioni agli interessi di una parte politica e che si rischiava di compromettere il libero esercizio del voto in Puglia, chiedendo che su queste situazioni vigilasse il Presidente della Repubblica, la domanda è: perché non ci hanno pensato prima e hanno fatto un irresponsabile ostruzionismo con emendamenti che non c'entravano nulla con la doppia preferenza.

il fatto è che non è stata applicata nel 2015 perché tutti i Gruppi politici erano sotto quella soglia, tranne il MoVimento 5 Stelle. Per questo approviamo questa legge oggi monca di questa parte, ma è il primo passo per rendere la Puglia migliore ed è per questo che dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

prendiamo atto. **Informativa del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento

Signor Presidente, onorevoli senatori, considero sempre la presenza in Parlamento un'opportunità per poter condividere la strategia che il Governo sta mettendo in campo sulla vicenda coronavirus e soprattutto un'occasione per poter ricevere spunti, idee e suggerimenti anche in vista delle prossime scelte che dovremo assumere da qui al 10 agosto. La dialettica democratica, anche se a volte aspra, sono convinto che renda il Paese più forte nell'affrontare un passaggio così difficile e anche per questo credo che non dobbiamo mai perdere di vista le ragioni di un confronto: qual è lo stato dell'arte? Come sta messa oggi l'Italia sul piano sanitario? In questa mia informativa vorrei partire da alcuni numeri che giudico molto rilevanti e che sono stati ufficializzati negli ultimi giorni dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), quindi dal principale istituto europeo che segue l'evoluzione dell'epidemia nel nostro continente. Questo centro ha indicato il tasso di incidenza su 100.000 abitanti negli ultimi quattordici in Italia il numero è pari a 5,7 casi, in Germania 8,4 casi, nel Regno Unito 12,6 casi, in Francia 19 casi, in Croazia 25,3 casi, in Spagna 53,6 casi, in Romania 75,1 casi. Sono numeri che credo spieghino meglio di tante altre parole il lavoro fatto in questi mesi e la situazione in cui si trova il in un contesto che è tutt'altro che semplice, perché nel mondo è sicuramente il momento più difficile. Procediamo a livello globale con circa un milione di nuovi casi a settimana, ci sono ormai 19 milioni di casi a livello globale e il numero dei decessi ha superato i 700.000. Sono numeri che non richiedono commento per la loro drammaticità e per la loro forza. Anche in Europa, nel nostro pezzo di mondo, la situazione è tutt'altro che tranquilla: basti guardare ai Balcani, dove i numeri sono assolutamente preoccupanti e in crescita e questo ci ha portato anche ad adottare alcune misure drastiche di contenimento, con divieto d'ingresso e di transito da alcuni di questi Paesi; la situazione è complicata anche in alcuni importantissimi Paesi europei. Voglio ricordare tra questi la Spagna, che nella giornata di ieri segnala quasi 1.800 casi,

Questo è un dato oggettivo che ci viene riconosciuto anche a livello internazionale. È un risultato di tutti. Voglio essere molto chiaro su questo punto: è un risultato è il risultato del Governo, è il risultato delle Regioni, è il risultato del Parlamento. È un risultato, prima di tutto, del nostro Servizio sanitario nazionale, di cui dobbiamo essere orgogliosi. *(Applausi)*. È un risultato dei nostri medici; è un risultato dei nostri infermieri; è un risultato dei nostri operatori sanitari, che hanno svolto un lavoro straordinario e ai quali, senza retorica, non smetteremo mai esprimere la nostra gratitudine. A questo proposito, permettetemi solo per un istante di ringraziare tutti i Gruppi parlamentari del Senato, proprio perché nella giornata di ieri si è consumato un voto importante ed è stata approvata la legge contro le aggressioni: una norma di grande civiltà, approvata all'unanimità alla Camera dei deputati e poi al Senato della Repubblica, che credo dia un segnale giusto, un segnale di un Paese che vuole prendersi cura di chi ogni giorno si prende cura di noi. Naturalmente questi risultati sono stati resi possibili dal comportamento dei nostri concittadini, che è stato straordinario e che dobbiamo ricordare in ogni passaggio. caso, una verità semplice: nessuno di noi, ad alcun livello, aveva un manuale di istruzioni. Siamo stati il primo Paese occidentale colpito dopo la Cina; non lo avevamo noi a Roma, non lo avevano i presidenti e gli assessori regionali nelle Regioni, non lo avevano i medici, gli infermieri, gli operatori negli ospedali. Eppure le istituzioni repubblicane hanno retto. Ecco, io penso che questa dovrebbe essere una valutazione condivisa della nostra comunità nazionale, del nostro Parlamento: le istituzioni repubblicane hanno retto. Basta tutto questo? È sufficiente? I dati che vediamo e quello che abbiamo fatto finora ci dicono che siamo al sicuro? Possono farci dire che la battaglia è definitivamente vinta? Io credo di no. La mia opinione è molto chiara e molto netta. Credo che stiamo molto meglio di come eravamo nei mesi di marzo, aprile e maggio e credo che l'Italia stia molto meglio rispetto a tanti altri Paesi del mondo e d'Europa,

che siamo fuori dalla tempesta - e questa è una verità - ma non siamo ancora in un porto sicuro. Abbiamo quindi bisogno di tenere ancora alto il livello di attenzione, di tenere alta la guardia, perché abbiamo recuperato tanto terreno ma ancora ci sono problemi, ci sono insidie, quindi serve la massima cautela. Dopo due mesi difficilissimi, quelli di marzo e di aprile in modo particolare, i due mesi del *lockdown*, come è noto abbiamo avviato, a partire dal 4 maggio, una lunga, graduale, prudente stagione di riaperture. Dobbiamo continuare esattamente su questa strada. Le prime riaperture, come ricorderete tutti, quelle del 4 maggio, hanno riguardato il cuore del nostro comparto produttivo: l'industria, la manifattura, l'edilizia, il commercio all'ingrosso. il 18 maggio - anche in questo caso lo ricorderete - abbiamo riavviato altre attività fondamentali del nostro Paese: penso ai servizi alla persona, alla ristorazione, ai bar. bar. Ancora, il 3 giugno abbiamo fatto un ulteriore passo, riaprendo i confini tra le Regioni e anche con tutti i Paesi europei. Insomma, è un percorso che un po' alla volta, con grande prudenza e gradualità, ci ha portato a una stagione di riapertura. Ad oggi, possiamo dare un giudizio positivo di questa prima fase di apertura. Eravamo preoccupati - senz'altro - perché nel momento in cui si riapre e in cui si riparte aumentano i contatti tra le persone e la possibilità di far ripartire il contagio. La mia opinione è che il sistema di monitoraggio che abbiamo costruito, e che in modo particolare l'Istituto superiore di sanità ha messo in campo insieme al Ministero della salute, in strettissimo coordinamento con le Regioni, ci ha consentito di valutare passo dopo passo l'impatto di queste riaperture. In realtà, i numeri ci dicono che la curva, nonostante le riaperture, almeno per una prima fase significativa ha continuato a piegarsi dal lato giusto. Ora, con la stessa chiarezza, i dati ci dicono che da qualche settimana siamo in una fase di sostanziale stabilità. Questo ci dice che ancora il virus circola, che ci sono *cluster* e focolai che spesso emergono nel nostro Paese, ma che il nostro sistema di monitoraggio e il sistema di prevenzione che abbiamo organizzato in ogni territorio ci mettono nelle condizioni di poter intervenire. Dovremo aumentare sempre di più la nostra capacità di resilienza, di essere veloci e rapidi, di poter immediatamente individuare questi focolai, isolare i casi positivi ed intervenire con grande determinazione quando questi si presentano. Penso che questo sistema di monitoraggio basato su ventuno criteri - su cui non torno - sia stato uno dei punti che ci ha consentito in questi mesi di gestire l'epidemia.

dal Ministero della salute, in collaborazione con l'Istat e con la Croce rossa italiana, che ringrazio per il lavoro straordinario che è stato messo in campo. Alla fine, abbiamo ottenuto una risposta positiva da oltre 65.000 persone: è il dato più alto a livello europeo; non c'è un'altra analisi sierologica fatta con un campione scientificamente affidabile (il nostro è stato costruito dall'Istituto nazionale di statistica). Questi primi dati che abbiamo ricavato, e che metteremo a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale, ci consentono di avere un'ulteriore fotografia di quello che è avvenuto in questi mesi. Anche in questo caso i numeri sono netti e chiari. Il 2,5 per cento delle persone del nostro Paese ha incontrato il virus e ha maturato nel proprio sangue gli anticorpi. È un numero che, proiettato su un valore assoluto, ci porta a un 1.482.000 persone. I dati di questa indagine sono molto dettagliati. Quello più significativo, che credo abbia una valenza più rilevante, riguarda la distinzione geografica: non è una sorpresa per noi, ma è del tutto evidente che c'è un enorme diversità nell'impatto che il virus e il contagio hanno avuto nelle diverse aree del nostro Paese.

cento). Invece, ci sono dati molto più bassi in altre Regioni. In modo particolare, voglio ricordare che nelle Regioni del Mezzogiorno c'è sempre una media che è sotto l'uno per cento (nessuna Regione del Sud raggiunge l'uno per cento), e le due isole sono addirittura allo 0,3 per cento. Questo dato ci dice che le misure attuate e il rigore delle misure messe in campo hanno consentito di fermare il virus dove era già arrivato in maniera molto significativa, cioè nelle aree geografiche dove l'impatto è stato più duro ed è arrivato in maniera anticipata sul piano temporale. Considerate anche un elemento che non ritengo irrilevante: la Spagna, l'altro grande Paese europeo che ha fatto un'indagine simile alla nostra, anche se con numeri leggermente ridotti, segnala segnala una percentuale di sieroprevalenza pari al 5 per cento. Noi siamo al 2,5 per cento ed anche questo è un dato che fa capire i termini di un impatto che c'è stato. stato. Sulla base delle valutazioni che ho fatto finora possiamo riaffermare quello che ritengo sia un fatto ormai evidente, cioè che non esiste un rischio zero e che siamo chiamati a continuare questo percorso di riapertura (perché noi continueremo ancora in questo percorso), nella nella piena consapevolezza delle cose che ho detto finora e, quindi, di questa linea di prudenza, saggezza e cautela che credo ci abbia positivamente portato fin qui. Quali sono le tre regole fondamentali che restano per noi decisive e che dobbiamo assolutamente mantenere nella fase che ci aspetta (nel mese di agosto e credo anche nella prima ripresa autunnale)? Si tratta di tre regole essenziali, riconosciute da tutta la comunità internazionale senza alcuna eccezione:

un metro; il lavaggio frequente delle mani. Sono tre regole comportamentali essenziali che dobbiamo provare assolutamente a consolidare ancora nel comportamento dei nostri concittadini.

queste tre regole, che devono essere patrimonio condiviso di tutto il Paese. Qui non c'è materia politica; su queste tre norme non c'è sinistra, destra o altro, in quanto si per continuare con prudenza un percorso di riapertura che io ritengo assolutamente indispensabile. L'ultima ordinanza che ho firmato nella giornata di sabato 1° agosto ripropone fondamentalmente queste tre regole essenziali. L'ordinanza è stata poi declinata sulla vicenda trasporti, ma è generica e ribadisce queste tre regole fondamentali che noi riporteremo anche come base essenziale del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È chiaro che altre attività apriranno; noi continuiamo questo percorso. Se siamo solidi su questi tre principi fondamentali e li condividiamo e se, in questa sintonia con il Paese, riusciamo a far vivere queste tre regole come

è quella di provare a far ripartire alcune delle attività che finora sono state sospese. Penso, per esempio, alle attività fieristiche (che sono di grande rilevanza per il nostro Paese) e alle

dei protocolli che il nostro Comitato tecnico-scientifico ha validato e messo in campo. Queste tre regole sono vincoli che provocano delle leggere restrizioni, ma è chiaro che se le paragoniamo alla fase di alla fase di *lockdown* che abbiamo vissuto, è del tutto evidente che siamo in una stagione diversa e che continuiamo a pagare un prezzo che ci mette però nelle condizioni di continuare questo percorso di riapertura dentro la stagione di convivenza con il virus. L'autunno sarà una stagione che dovremo affrontare con queste regole e con la massima accortezza. Mi piace ricordare in quest'Aula del Senato, dove mi era stato richiesto in modo particolare da un'interrogazione del senatore Romeo e degli altri senatori del Gruppo della Lega Nord, che in queste ore

l'orizzonte con cui affrontare la fase della ripresa. Era una richiesta arrivata da questo Parlamento cui mi ero impegnato a rispondere positivamente e mi fa piacere, oggi, poter dare questa informazione.

Credo molto in questo rapporto positivo, nel rispetto delle reciproche differenze e delle reciproche autonomie. Non vi è dubbio che sia la politica a dover scegliere, ma sono profondamente convinto che la politica possa scegliere meglio se ha - diciamo così - la capacità di ascolto, di dialogo e di comprensione dell'evidenza scientifica che può arrivarci quotidianamente dai nostri scienziati. Penso che la politica sia più forte, quindi permettetemi di dire che il lavoro del Comitato tecnico scientifico, anche su questo piano, sui protocolli di sicurezza che stiamo costruendo, è molto importante e anche in questo caso permettetemi di usare questa informativa per affermare che il dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio ha già provveduto a consegnare i verbali a chi ne ha fatto richiesta e che continueremo esattamente su questa linea. *(Applausi)*. La trasparenza è stata, per quanto mi riguarda, fin dall'inizio una regola fondamentale che ci siamo dati

luogo, la scuola è stata oggetto di numerosi dibattiti e ho avuto modo di dire che riterremo il *lockdown* definitivamente chiuso nel nostro Paese solo nel giorno in cui tutte le scuole di ogni ordine e grado, senza differenze e senza distinguo, potranno riaprire. Chiudere le scuole è stata, per quanto mi riguarda anche sul piano personale, la scelta più difficile da fare. Purtroppo è stata una scelta indispensabile. Anch'essa spiega i numeri di cui ho provato a ragionare e le differenze tra noi ed altri Paesi d'Europa e del mondo, però è evidente che a settembre dovremo ripartire. Confermo che l'intenzione del Governo è molto chiara su questo punto: le scuole riapriranno e riapriranno tutte. Il nostro obiettivo è che riaprano in piena sicurezza. Stamattina è stato firmato il protocollo di sicurezza tra il Ministro dell'istruzione e le forze sociali e riteniamo che questo sia un altro passo avanti in questo percorso. Sulle scuole stiamo lavorando per ripristinare una relazione più organica tra l'universo della salute e l'universo della scuola. Tale relazione organica strutturata è esistita nella storia del nostro Paese. Nel 1961 fu approvata una norma che introduceva nel nostro ordinamento la medicina scolastica. Tale norma si è persa negli anni Novanta, in una stagione di tagli, una stagione di austerità in cui la contrazione della spesa pubblica ha avuto l'effetto, probabilmente, di rompere questo legame. Ora, io non penso che dobbiamo tornare esattamente ad un modello del passato, ma il tema di fondo di una relazione organica, non episodica, strutturata tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie dei nostri distretti e i plessi scolastici e gli istituti sia particolarmente importante e lo sia in modo particolare in questo momento, perché noi non dobbiamo lasciare soli i nostri insegnanti e i nostri presidi. Se c'è una questione che è di natura sanitaria, c'è bisogno che chi ha la competenza in tale ambito dia una mano e stia al fianco dei nostri presidi e dei nostri insegnanti per gestire la vicenda.

battaglia, una sfida in cui il nostro Paese è convintamente inserito e che io ritengo particolarmente strategica. La mia opinione è che un vaccino sicuro, un vaccino sicuro, certo e chiaramente validato con tutti i canoni scientifici possa metterci nelle condizioni di vincere definitivamente questa battaglia. Il nostro Paese sta investendo con tutte le energie di cui dispone in una sfida che, come è ovvio, non è la sfida di un Paese, non è la sfida di un continente ma è la sfida di tutto il mondo in questo momento. Vi ho già informato dell'alleanza per i vaccini, che l'Italia ha sottoscritto con Francia, Germania e Olanda. Questa alleanza ha rappresentato il motore dell'iniziativa sui vaccini della Commissione europea. Noi abbiamo sottoscritto un primo accordo molto importante con Astrazeneca. Chiaramente, oggi stiamo parlando di un candidato vaccino, ma tale accordo ci consentirà di avere, se questo candidato vaccino dovesse superare tutte le prove, le prime dosi già entro la fine del 2020. Questo candidato vaccino, che oggi sembra essere quello più avanti in termini di tempo, è un candidato vaccino che è stato studiato, elaborato e progettato presso l'Università di Oxford. Voglio, però, ricordare che il vettore virale, che è un pezzo fondamentale di questo impianto, viene prodotto presso l'azienda Irbm di Pomezia. Quindi, c'è anche un pezzo del nostro Paese. E l'infialamento di questo stesso vaccino, prodotto da Astrazeneca, avverrà, per tutte le dosi europee, presso la sede della Catalent di Anagni.

Stiamo parlando di un candidato vaccino. Anche se abbiamo un contratto che dice che esso arriverà, se andrà bene, già alla fine dell'anno, è però ancora un candidato vaccino. La rivista *Lancet*, che è una delle principali riviste scientifiche sul piano internazionale, ha riportato uno studio sulla fase 1 e 2 di questo vaccino Astrazeneca Oxford-Anagni Pomezia, secondo il quale, sostanzialmente, la fase 1 e 2 hanno avuto risultati molto incoraggianti. La fase 3, che è in corso, è una fase che avrebbe dovuto essere fatta da tutti in Europa. Quando, però, la curva del contagio in Europa si è abbassata, è stata spostata in Brasile, in Sudafrica e in altre parti del mondo. Il nostro auspicio è che possano, nel più breve tempo possibile, arrivare notizie incoraggianti quanto quelle che sono già state diffuse dalla rivista *Lancet*. Ancora sui vaccini. Oltre ad Astrazeneca, con la Commissione Europea stiamo lavorando per chiudere contratti con tutte le altre grandi case farmaceutiche che sono è un gruppo ristretto della Commissione europea e l'Italia è all'interno di questo gruppo ristretto proprio perché fa parte della prima alleanza dei vaccini con Germania, Francia e Olanda. Noi proveremo, nelle prossime ore, a livello di Commissione europea, a chiudere ancora tanti contratti, perché, appena una di queste compagnie dovesse darci una notizia positiva, saremo nelle condizioni di poter usufruire immediatamente del vaccino nel nostro Paese.

del Lazio, una realtà del nostro Paese, anch'essa importante. In questo caso, la fase di sperimentazione *in vitro* e sugli animali si è completata ed è iniziata la fase di sperimentazione sull'uomo, che avverrà all'istituto Spallanzani di Roma e al Policlinico Rossi di Verona.

è una risposta all'interrogazione n. 3-01834, presentata in questa Aula dal Gruppo Fratelli d'Italia. Come sapete, i mesi del Covid-19 sono stati mesi difficili per tutte le altre patologie. Per tre mesi il Paese è stato concentrato quasi esclusivamente sul Covid-19 e le nostre strutture sanitarie, ospedaliere e non, hanno concentrato la stragrande maggioranza delle proprie energie per fronteggiare questo nemico, che è stato il nostro principale avversario. Si trattava di salvare vite e non poteva che essere così. La conseguenza è che tutta una serie di prestazioni sono state sospese, sono state rinviate, e noi ci troviamo in una situazione in cui già avevamo un peso significativo in termini di liste di attesa e ora, purtroppo, col passare delle settimane, questo peso è diventato Ho proposto al Governo, in modo particolare al Ministro dell'economia e delle finanze, che in questo decreto si possano individuare risorse, pari a mezzo miliardo di euro, per quel piano straordinario, che veniva richiesto nell'interrogazione di Fratelli d'Italia e che ritengo sia molto utile e importante: mezzo miliardo perché il nostro Servizio sanitario nazionale possa, nei prossimi mesi, recuperare le visite mediche, gli *screening*, gli interventi chirurgici e le prestazioni diagnostiche, che in queste settimane di Covid-19 non siamo riusciti purtroppo ad affrontare. Credo che anche questa sia una notizia positiva *(Applausi)*, che va nella direzione giusta e che testimonia l'impegno del Governo e del Parlamento in questa situazione. *(Applausi)*.

che ci dividono ma che ci appartengono, perché veniamo da lontano, riesce difficile non approvare e non apprezzare il suo taglio, il suo piglio, il suo modo di impostare il ragionamento, rispetto a un Governo che

questo suo modo di approcciare il Parlamento. gli amici spagnoli sono nel pieno della bufera, che noi abbiamo vissuto qualche mese fa. Evidentemente questo non ci rassicura, nel momento in cui andiamo ad aprire la stagione estiva, il turismo e le frontiere, che naturalmente sono permeabili e devono esserlo. Signor Ministro, lei ci riferisce di un costante sistema di Il sistema di monitoraggio a cui fa riferimento è ancora, purtroppo, un sistema che insegue i sintomi e la manifestazione febbrile. Lei sa bene che, se non c'è la manifestazione febbrile, il tampone generalmente non viene fatto. Quindi ancora siamo nella prima fase, nel primo livello di

ci riferisce essere stata utile: a mio avviso è stato invece un esercizio semplicemente statistico, tanto che addirittura anche l'Istat poneva la soglia dei 150.000

però ricordiamo anche i tre pilastri che ci suggerisce quell'Organizzazione abbastanza inutile, ma che su questo potrebbe risultare invece coerente, ossia il tracciamento, il trattamento

l'indagine di sieroprevalenza a mio e nostro avviso non è stata ampiamente all'altezza delle premesse e soprattutto dei costi; l'*app* Immuni

un sistema di protezione per il personale medico-sanitario e per quello scolastico rispetto alla possibilità che ci sia un problema di natura penale.

- che, oltre ad essere la mia Regione, è la più piccola e quindi ci aiuta a descrivere meglio il problema - è stato quantificato il ritardo: la popolazione in lista d'attesa è pari a metà

con la messa a disposizione di danaro, ma il Governo si deve far carico anche di dettare alcune regole per, ad esempio, un diverso coinvolgimento del privato. Ci sono Regioni che sulla diagnostica tengono il privato ancora a circa

Concludo ringraziandola per il modo con cui lei approccia, ma raccomandandole, come fin dall'inizio ho fatto, un ruolo maggiormente da protagonista nell'azione del Governo per tutto ciò che sta accadendo e accadrà nei prossimi mesi. *(Applausi).*

dialogare con il Parlamento e il Senato sui prossimi provvedimenti che il Governo assumerà da qui al 10 agosto. Siamo contenti perché, pure in questa situazione così complicata, stamattina ci ha portato delle buone notizie, a partire dalla trasparenza dei tecnico-scientifico (CTS). Non più tardi di ieri abbiamo avuto una discussione in Assemblea a questo proposito e siamo molto contenti che questa questione è stata sbloccata all'insegna della trasparenza

e Istituto superiore di sanità, sta avendo dei frutti sui quali possiamo costruire le politiche successive. Ne abbiamo parlato tanto quando il Senato ha approvato il

come su questa base possiamo fondare le nostre politiche, a partire dai dati sugli asintomatici e su chi ha sviluppato anticorpi. È, quindi, essenziale. I dati che lei riportava all'inizio del suo discorso rispetto all'Unione europea naturalmente ci confortano. confortano. Ci devono far usare tutte le accortezze se i Paesi intorno hanno un numero più alto di contagiati. Dobbiamo avere molta accortezza su questo. Ci dicono che noi abbiamo fatto, come lei ricordava, in Italia un *lockdown* molto serio e rigoroso. Ringrazio i nostri

ospedaliera degli Spedali Civili di Brescia domenica scorsa - una struttura che è stata particolarmente colpita - dove ho potuto constatare con mano quello che i medici, gli infermieri, il personale ausiliario, gli addetti alle pulizie negli ospedali hanno compiuto, con quanto sacrificio e abnegazione. soprattutto quanta competenza, informazioni ed esperienza sul campo hanno accumulato

la professionalità del nostro sistema sanitario è in grado ora anche di trasferire esperienze non solo nell'ambito del territorio nazionale, ma su base mondiale. Condivido pienamente le sue parole sulla prudenza,

Lei parlava di sintonia con le cittadine e i cittadini italiani: tutti noi politici dobbiamo fare uno sforzo enorme; non ci sono colori politici su questo - condivido pienamente perché possiamo essere in sintonia con il popolo italiano per infondere il rispetto, la responsabilità di queste tre regole: mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani. Dobbiamo fare tutti uno sforzo direi educativo rispetto a questo tema nei messaggi che mandiamo e nei comportamenti che assumiamo per trasferire soprattutto ai nostri giovani

In questa fase, per tenere insieme i tre nodi (prudenza, convivenza e riapertura) dobbiamo tenere insieme salute, lavoro, scuola e trasporti. Qual è oggi il compito della politica a mio avviso? Fare in modo che la convivenza con il virus in questa fase non porti al risultato di creare ulteriori disuguaglianze nel nostro Paese.

pensoche il Governo debba agire con una relazione organica e in sintonia perché non ci sia produzione di disuguaglianze rispetto a chi non può. Infatti, chi non riuscirà a spostarsi in maniera agevole, potrà usufruire di mezzi privati, e in questo senso ritengo che compito della politica sia attenzionare e monitorare anche il piano di trasporti che nei vari territori del nostro Paese

dobbiamo far vivere questo provvedimento e attrezzarci, perché più la popolazione è tranquilla,

Un'attenzione particolare - lo ricordiamo sempre - merita la questione delle famiglie con disabilità, Ministro, perché ci sono ancora tantissimi problemi di apertura dei centri diurni, residenziali e semiresidenziali: questo è un tema fondamentale. fondamentale. Se in questa fase così delicata agiamo con responsabilità tutti insieme, ce la possiamo fare ad uscire da questa brutta epidemia

all'altezza della serietà e della responsabilità dei cittadini durante il *lockdown* e andare avanti in questo percorso.

non solo il suo stile, ma la qualità del suo lavoro e del Governo. Abbiamo già avuto modo di sottolineare più volte quanto condividiamo questo impegno nella convivenza con il virus, che richiede prudenza ed intelligenza,

Ne avevamo parlato, Ministro, ed è un punto importante: stiamo parlando di filiere economiche importanti, nella misura in cui giustamente ciò avviene attraverso i protocolli che il CTS ha approvato. Apprezziamo anche la scelta di pubblicare i verbali

si poteva evitare il siparietto di ieri, ma questo è un altro discorso e vale per tutti: vale per chi l'ha fatto e vale per chi ha causato quel siparietto. solo porre due problemi: il primo è il rafforzamento della cooperazione con le Regioni. Il Presidente della Repubblica ha detto una cosa che condivido moltissimo, parlando della leale collaborazione. Da questo punto di vista la vicenda dei treni deve

molto importante che, alla ripresa, tutti dovremo portare avanti, in riferimento al piano di investimenti,

e voglio dirlo con molta chiarezza, perché ci sono dei nodi politici che vanno affrontati. fare attenzione a non pensare di affrontare la questione delle liste d'attesa con un processo ancora più significativo di esternalizzazione, questo produrrebbe un problema relativo alla qualità, alle professionalità e alle prospettive del Sistema sanitario nazionale pubblico, che è stato l'unica vera garanzia che abbiamo avuto nella lotta al Covid. È bene, colleghi, che queste tematiche riusciamo a discuterle in modo esplicito e chiaro. Anche in quest'Aula, signor Ministro, ho già avuto modo di chiedere un momento di discussione strategico sulla sanità, che sarebbe molto importante. Questa Assemblea mi sembra matura per poter svolgere questa discussione e per poter sciogliere insieme dei nodi che abbiamo davanti e che avevamo davanti anche prima del Covid-19 e che il Covid ha, da questo punto di vista,

Apprezzo quanto lei ci ha detto oggi e devo dire che molte delle cose che ha riferito le avevamo già sentite, perché anche l'articolo sul «New York Times» cita l'Italia come modello a livello internazionale. Credo che questa sia una soddisfazione importante per il nostro Paese, per il nostro Governo

quindi le diamo atto di una fiducia ulteriore. Secondo i dati che stanno circolando, purtroppo siamo davvero contornati da Paesi che riteniamo alla nostra altezza, come Germania, Francia e Spagna,

la mascherina sta diventando lo stesso: quando esco di casa, la prima cosa che mi viene in mente è chiedermi se ho la mascherina

per tutti questi mesi. Dobbiamo dare atto che hanno bisogno di avere relazioni interpersonali dirette. La teledidattica può essere un aiuto, ma non è sicuramente la scuola che noi vogliamo. Ovviamente occorre un'interazione maggiore con le Regioni, perché sono quelle che se ne dovranno occupare. La collega parlava prima del trasporto: i trasporti scolastici sono a carico delle Regioni, come sono a carico degli enti locali. Serve quindi un'interazione maggiore fra questi enti e ovviamente serviranno fondi (ma ne metteremo a disposizione).

il ruolo e i toni, se mi posso permettere, che ci portano a pensare bene di lei. Questo è un complimento che io le rivolgo, mi creda, con sincerità (a parte che non so dire bugie e questo è uno dei miei noti difetti, da politico, perché si dice che invece di solito i politici dicano

è l'esatta rappresentazione di quel che lei vede. Lei, signor Ministro, si sta guardando intorno e vede sostanzialmente i banchi del Senato vuoti. è la dimostrazione di quanto sia del tutto inefficace, da un punto di vista squisitamente, e non tecnicamente, parlamentare, la funzione dell'informativa il Ministro deve dare ai sensi dei provvedimenti collegati al decreto-legge n. 19, nei quali si decise, per cercare di ridare centralità al Parlamento, un pannicello caldo. A noi fa piacere ascoltarla e ci fa piacere avere notizie sullo stato dell'arte, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria, tra l'altro prolungata fino a fine ottobre.

centrale il problema del rapporto tra Governo e Parlamento, tra potere esecutivo e potere legislativo. Il ruolo del Parlamento è purtroppo del tutto sminuito in questa fase; è assolutamente inefficace ed incongruo. Lei ci viene a dare delle notizie, che potrebbe dare anche, come faceva il presidente Conte nel periodo del *lockdown*, attraverso delle conferenze stampa rivolgendosi direttamente ai cittadini italiani e non quindi

Ministro, visto che lei proviene da un partito di sinistra che crede nella divisione dei poteri, nella centralità del Parlamento e nella funzione della politica, soprattutto della politica rappresentativa, quella parlamentare, questo deve per forza di cose metterla a disagio. Di fatto, siamo qui soltanto ad ascoltarla; ognuno di noi parla - abbiamo dieci minuti per Gruppo per esporre le nostre opinioni - ma il problema resta questo. È in corso, È in corso, come è noto, un *referendum* che attiene ad una decisione suicida di questo Parlamento, cioè quella di tagliare quasi la metà dei parlamentari italiani, riducendolo sostanzialmente a un

Però anche questo nasce da un'evidente esigenza, ossia ridurre il Parlamento a cosa di poco conto. Signor Ministro, faccia caso a quello che sta accadendo dal *lockdown* ad oggi.

abbiamo contenuto i danni nel nostro Paese e che oggi, sulla base delle indicazioni che le sono state conferite, anche attraverso il tasso di incidenza di cui ci ha parlato, siamo messi meglio di altri Paesi dell'Unione europea. ammettere (lo ha anche detto) che non siamo fuori dal pericolo, che c'è un problema di Covid tutt'ora presente, che probabilmente avremo problemi anche durante l'autunno e che quindi, per queste ragioni, bisogna mantenere assolutamente le tre regole sull'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, sul distanziamento di un metro e sul lavaggio delle mani. Benissimo, lo faremo. Tutto questo, però, contrasta con un atteggiamento contraddittorio, perché se è vero quello che lei ci ha detto, ci deve allora spiegare per quale benedetta ragione il suo Governo ha stabilito che un *referendum* che coinvolgerà

Concludo dicendole: non dimentichi che lei, da Ministro della salute, ha giustamente, correttamente a mio sommesso avviso, bloccato i collegamenti con 16 Paesi

Ne prendiamo atto. È vero che siamo, per qualcuno, già con la valigia in mano e pronti per andare in vacanza, però questi sono temi ai quali ci dobbiamo abituare e soprattutto ai quali dobbiamo dare la necessaria importanza.

Premetto che ci piacerebbe anche condividerne il contenuto, quindi non solo sapere che ha tenuto conto della nostra indicazione. È certamente vero che il suo operato è all'interno di un campo minato perché il Governo sta lavorando con un'approssimazione che ci preoccupa,

con la questione dei banchi che ormai è diventata veramente oggetto addirittura di barzellette, o dal Presidente Conte, più impegnato a gestire il rinnovo e il procrastinarsi dei Servizi segreti piuttosto che a dare l'attenzione che deve al Parlamento. Oppure pensi alla sua collega Lamorgese che oggettivamente sta dando la pessima prova di un Ministro "colabrodo" che non riesce a gestire l'ordine pubblico e la sicurezza sul territorio nazionale, nemmeno ai confini. Che dire poi della sua collega De Micheli con cui abbiamo visto che non siete esattamente allineati quando c'è da definire come si va in treno, in aereo o come ci si sposta da una parte all'altra. *(Applausi)*. Questa è la squadra di Governo, Ministro. Questa è la sua squadra di Governo, quindi non ne abbia male se poi siamo anche abbastanza in disappunto rispetto a quanto sta avvenendo perché, ribadisco, se lei viene qui e ci rassicura, quello che fa la squadra di Governo è ben altra cosa. Il suo intervento è stato rassicurante, come è giusto che sia, ma ci deve essere anche una relazione con la realtà. Questa relazione manca, lo vediamo costantemente, come dicevo prima, con l'attività del Governo intero. E poi ci sono dei quesiti che vogliamo porre e su cui vogliamo delle risposte. Abbiamo saputo che dei 150.000 kit per i test sierologici previsti,

Lampedusa. Lei è stato lì dentro? Se non c'è stato ci vada. Vada a vedere che cosa accade lì dentro e quali rischi per la salute delle persone ci sono. Oltretutto, il suo collega

Quanto ai positivi stranieri, salvati al mare, vengono tutti sottoposti a test e tamponi e molti di loro ripartono immediatamente». Bontà di Dio: il 25 per cento si applica su 15.000, dall'altra parte ci sono 60 milioni di Italiani. Ma che stiamo dicendo? Ma almeno sappiamo

Ed è inaccettabile ancora di più se messo in relazione alla grande fatica e al grande sforzo al quale si sono sottoposti i cittadini italiani e gli stranieri regolari presenti sul nostro territorio rispettando le regole.

Noi ci stiamo opponendo e si oppongono i cittadini di quel territorio, perché non è ammissibile che, quando un Governo non riesce a garantire che chi viene messo in quarantena ci resti, addirittura crei ammassamenti di centinaia di potenziali contagiati semplicemente perché non sa dove metterli. Questa non è una gestione seria, signor Ministro, e se non riguarda il suo Dicastero se ne faccia carico, perché l'attività del Governo riguarda tutti gli italiani. E se il ministro Lamorgese non è in grado di fare il proprio dovere, il Governo se ne deve prendere carico! Signor Ministro, veniamo poi alla nota questione del segreto di Stato imposto sui verbali del comitato tecnico scientifico. Lei oggi viene qui in Aula e, riporto testualmente, ci dice che: «la trasparenza è sempre stata la scelta del Governo». Non mi pare. Avete posto voi il segreto. Quando la Fondazione Einaudi ha chiesto la disponibilità dei verbali, avete opposto voi il segreto, ricorrendo in Consiglio di Stato. E se lo avete fatto è perché non volevate che fossero messe a disposizione informazioni per i cittadini italiani, dicendo testualmente, come ha detto l'Avvocatura dello Stato: «Perché si rischia pregiudizio per la sicurezza pubblica». Ma di che stiamo parlando? Voi oggi siete arrivati a togliere il segreto di Stato solo su una parte. Andando, infatti, a consultare la parte oggi già disponibile, vediamo che vi sono 3577 pagine di allegati non messe a disposizione. *(Applausi)*. Il primo verbale parte dal numero 12, mentre sappiamo benissimo che lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Governo il 31 gennaio e la costituzione del Comitato tecnico-scientifico risale al 5 febbraio. Signor Ministro, la trasparenza la si fa dalla A alla Z. Se poi lei questa situazione l'ha subita e non la condivide, è un problema suo e lo affronterà con il resto del Consiglio dei ministri. Io dico, però, a chi voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, che l'avete chiuso e l'avete sigillato proprio bene. E se ieri, qui in Aula, non avessimo preso noi posizione, quella scatoletta di tonno sarebbe, addirittura, ancora chiusa a chiave Questa non è trasparenza: questo è creare opacità e preoccupazione nei cittadini su quali siano le vere finalità che stanno dietro alla gestione dell'emergenza sanitaria così come proposta dal Governo. Governo. Il dubbio, infatti, viene. Tornando, però, a quanto dicevo all'inizio, signor Presidente, ci preoccupa l'approssimazione nella definizione delle regole e delle azioni da parte del Governo, a partire dalla scuola, con quella ridicola scelta scelta di sostituire i banchi fissi con quelle cose con le rotelle, che chiamano banchi mobili ma che sono, brutalmente, delle sedie a rotelle con la ribaltina. Una cosa orribile, sulla quale non so neanche come potremo formare i nostri giovani

della scuola, che è stata eradicata ed estirpata ormai da anni dalla scuola e che, invece, lì dentro deve ritornare. In questi tempi, ancora di più la presenza di presidi medici seri, costantemente presenti a monitorare l'andamento delle scuole e di un possibile contagio, è fondamentale per impedire che si interrompano ancora una volta gli esami piuttosto che le sessioni di istruzione. Non servivano gli scienziati per dire questo, serviva semplicemente la capacità politica di amministrare, serviva guardare avanti da quando la crisi è iniziata, sapendo bene che la scuola deve riaprire.

prevedendo quindi tempi abbondantemente lunghi, dico che ora è necessario dare garanzie agli italiani anche in merito ad una seria campagna vaccinale antinfluenzale.

Di questo abbiamo certezza: se non si faranno azioni di questo tipo, arriveremo veramente ad avere una grave crisi, e non ci saranno più le scuse dell'improvvisazione iniziale, perché questo non ci era mai capitato, ma ci troveremo di fronte a una sciagura prevista. Concludendo, vogliamo impegni seri. Non vogliamo semplicemente una lenzuolata di impegni presi qui dentro all'inizio di agosto, quando tutti hanno ormai le valigie pronte per andare in vacanza e lo dico ancora ai senatori del PD, totalmente assenti. abbiamo la preoccupazione che la gestione da parte del Governo, come è stata prospettata fino ad adesso, sia essenzialmente improntata a manipolare il consenso dei cittadini, creando ad arte delle preoccupazioni e dando poi delle soluzioni. Questa non è una gestione seria. Siamo molto preoccupati, perché il nostro è un Paese che ha saputo gestire, per la grande responsabilità degli italiani, questa situazione di crisi, ma non può essere gettato nel panico per la sottovalutazione dei problemi che ci troveremo questo autunno.

come ha correttamente ricordato poc'anzi il Ministro della salute, sebbene il *trend* epidemiologico attuale non raggiunga i livelli di criticità dei mesi scorsi, in questi giorni in questi giorni tuttavia si registra un lieve, ma costante aumento dei casi di contagio. Il bollettino del Ministero della Salute del 5 agosto rilevava che nelle ultime ventiquattro ore vi era stato un aumento dei nuovi contagi, cioè 384 casi a fronte dei 190 del giorno precedente, e purtroppo anche dei morti, arrivati a 10 rispetto ai 5 del giorno precedente. Questo momento deve essere quindi interpretato come monito assoluto a non allentare le misure e a porre in essere i corretti presupposti per interventi tempestivi ed efficaci, nell'infausta ipotesi di una ripresa dell'epidemia. In verità la situazione è molto più seria nel resto del mondo, se se guardiamo a ciò che sta avvenendo nei Balcani o alla recrudescenza dell'epidemia in Paesi come la Spagna, la Francia, la Germania o, ancora, alla fase molto complessa che stanno vivendo gli Stati Uniti,

non può essere assolutamente abbassata e riteniamo assolutamente giuste e sensate le scelte adottate dal Governo, fondate su un razionale di evidenze e di precise valutazioni tecniche. Sotto il profilo sanitario, difatti, sebbene la curva epidemiologica dei contagi si sia abbassata e rimanga stabile da qualche giorno, i dati che si registrano dimostrano che il virus continua a circolare ancora, dando vita a circoscritti focolai, che senza adeguate misure e cautele potrebbero alimentare una ripresa dell'epidemia. Questa situazione si può paragonare a quella di un incendio che è stato domato, ma che non è stato ancora del tutto spento, perché piccoli focolai covano sotto la cenere,

In ogni caso, il virus non può e non deve considerarsi un nemico lontano e passato: è ancora presente e, se non viene tempestivamente circoscritto e arginato, l'infezione rischia di crescere nuovamente e accelerare. Lei, signor Ministro, ha fatto bene a ricordare - e sarebbe bene che lo facessimo più spesso - che ancora non abbiamo vaccini né farmaci in grado di distruggerlo o contrastarlo: non abbiamo alcuna arma efficace che non sia la prevenzione del contagio, che si può attuare attenendosi a precise norme, come appunto il rispetto della distanza interpersonale, l'uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani. Come rilevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue ultime comunicazioni a quest'Assemblea, la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria affinché le decisioni assunte con i decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020 non perdano efficacia e perché le misure vigenti, approntate con lo stato d'emergenza, continuino ad avere copertura normativa. Cautela, prudenza e rispetto delle norme per la tutela della nostra salute devono essere le parole d'ordine. Pochi giorni addietro il signor Presidente della Repubblica ha detto: "Non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà. Naturalmente occorre tener conto anche del dovere di equilibrio con il valore della vita, evitando di confondere la libertà con il diritto di far ammalare altri". La proroga non significa un altro blocco di tutto il Paese o una limitazione della libertà dei cittadini, ma ha lo scopo di mantenere le condizioni per riprendere gradualmente una vita sociale, economica e produttiva normale, secondo criteri di sicurezza, nel rispetto delle libertà di tutti. di tutti. Sarebbe opportuno pertanto che in queste circostanze ancora straordinarie l'azione di Governo fosse sostenuta da tutti, dalle Regioni e anche dalle opposizioni, le quali ultime, a parere del sottoscritto, potrebbero evitare talune critiche improvvide, talvolta anche infondate, che generano solo confusione nella popolazione e nulla hanno a che vedere con l'obiettivo primario dell'azione di questo Governo, costituito dalla tutela della salute e della libertà di tutti i cittadini. Chiudo il mio intervento citando alcune delle parole con le quali l'Italia è stata apprezzata a livello internazionale per la gestione dell'emergenza, dopo lo scoppio

eravamo un posto da evitare in tutti i modi e un epicentro da incubo; oggi siamo un modello, seppur non ancora perfetto, di contenimento del virus, perché siamo stati in grado di dare lezioni al resto del mondo, ai nostri vicini e agli Stati Uniti, grazie alle azioni e ai provvedimenti adottati da questo Governo. Non vanifichiamo quindi quanto fatto sino ad oggi: grazie, signor Ministro, Governo

settantacinque anni dalla mattina in cui l'Aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Tre giorni dopo sarebbe toccato a Nagasaki: stesso ordigno e stesso scenario di morte e devastazione. Credo sia nostro preciso dovere oggi rendere omaggio alle migliaia di vittime provocate da quegli attacchi. Ma ancor più credo sia un nostro preciso dovere rinnovare l'impegno affinché le armi nucleari vengano messe al bando, così come prevede il trattato dell'ONU

Voglio condividere con voi l'*incipit* dell'articolo 11 della nostra Carta costituzionale, che ci dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Sono parole che esprimono un principio assoluto, ma anche un'intrinseca necessità di agire. Escludere la guerra non significa automaticamente promuovere una politica di pace. Viviamo in un tempo in cui la questione del riarmo nucleare è tornata di grandissima attualità c'è un ritorno di interesse, oltre un *escalation* di conflitti, tra le maggiori potenze. Attualmente la violenza è sempre più accettata come metodo di risoluzione dei conflitti non soltanto tra i diversi Stati. Non possiamo e non dobbiamo essere spettatori. Non dobbiamo rimanere indifferenti. Gli studiosi parlano di nuova era del rischio, che non è stato mai così alto, neppure agli inizi degli anni Cinquanta, quando USA e URSS si fronteggiavano con i primi ordigni all'idrogeno. La recente svolta nella geopolitica delle armi atomiche ha condotto il metaforico orologio dell'apocalisse, ideato dagli scienziati dall'università di Chicago, a cento secondi dall'ora «x». Cento Cento secondi sono poco più di un battito di ciglia, che a me riportano alla mente una delle tante testimonianze offerte all'opinione pubblica dai sopravvissuti dei bombardamenti in Giappone: risale a una decina di anni fa e appartiene a una donna che il giorno dell'atomica a Hiroshima era solamente una bambina. Già allora lei ci implorava di rendere forte la voce di chi poteva dar conto dell'orrore e ci avvertiva: se l'umanità non eliminerà le armi nucleari, le armi nucleari

due o tre mesi fa la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha spiccato 126 ordini di custodia cautelare

presso quell'ospedale, uno dei più grandi della Campania, si era installata una sede sociale - queste sono le parole che usa il testo della ordinanza della procura della procura - dell'alleanza di Secondigliano, il cartello camorristico nel quale sono confluite le tre più potenti e temibili

Avevano anche allestito una fabbrica di certificati falsi per truffe sistematiche alle compagnie di assicurazione. Alcuni pentiti hanno poi dichiarato che questa diffusa infiltrazione era comune anche agli altri grandi ospedali napoletani, tant'è che le inchieste sono in corso a macchia d'olio.

La commissione d'accesso - stando alle notizie di stampa - ha redatto un'articolata e puntuale relazione, in piena coincidenza con i contenuti e le valutazioni della procura della Repubblica di Napoli. Dopodiché, il prefetto di Napoli, sulla base di tale relazione - stando sempre a riferimenti di stampa - ha avanzato la proposta di commissariamento della ASL Napoli 1 per infiltrazioni camorristiche. La proposta è da diverso tempo nelle mani del Ministro dell'interno, che, però, non conclude il procedimento, e questa è la ragione per la quale ho preso la parola, signor Presidente. conclusione, qui c'è anzitutto un problema di diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione come diritto fondamentale del cittadino e interesse primario della collettività: l'unica volta che la Costituzione, con riguardo a tutti i diritti soggettivi, contrassegna un diritto con l'aggettivo "fondamentale", e questo la dice lunga per quanto riguarda la gerarchia dei valori. Di più, c'è la grave compromissione dell'ordine pubblico (ex articolo 117, secondo comma, lettera h), dalla Costituzione). C'è quindi un'esigenza di legalità e di trasparenza. Non è possibile che il Ministro dell'interno non decida e temporeggi,

di attivare i meccanismi sollecitatori previsti dal Regolamento del Senato affinché ci sia una pronta risposta, che è attesa non soltanto da noi senatori interroganti, ma da tutta la comunità.

su finanziamento pubblico. Sono in 293. Hanno sempre dato problemi di ordine pubblico. Alcuni vivono in maniera *borderline*, altri sono dei veri e propri delinquenti, a questo si è aggiunto un altro problema. Grazie all'opera di monitoraggio anti-Covid della Regione Veneto, di questi 293, stamattina 136 risultano positivi al Covid. Queste persone rifiutano la quarantena, rifiutano il distanziamento così come l'uso delle mascherine, portando problemi che si intrecciano tra ordine pubblico ed emergenza sanitaria, con un dispiego di Forze dell'ordine costante.

Il problema è gravissimo, che arreca danni anche alle comunità locali. Ho sentito i sindaci Mario Conte di Treviso e Renzo Carraretto di Casier che sono in allarme.

come già chiesto dalle amministrazioni della Regione, della Provincia e dei Comuni coinvolti. In merito alla seconda: lo Stato italiano dia seguito alle domande di risarcimento danni presentate dai due sindaci di Treviso e Casier, Conte e Carraretto,

seguente: non pretendo - e mi rivolgo in particolare alla parte più sinistra di questa maggioranza - che imitiate o impariate da quello che ha fatto il ministro Salvini, perché siete impermeabili alla conoscenza. Abbiate, però, almeno un po' di compassione nei

il 6 agosto del 1863 il 6 agosto del 1863 a Pietrarsa, Portici, presso un'eccellenza dell'industria del Sud, con circa 1.200 lavoratori, di cui 800 specializzati. L'eccellenza era l'opificio borbonico voluto da Ferdinando II di Borbone, azienda poi ceduta e caduta in rovina dopo la fine del Regno delle due Sicilie; la fabbrica venne privatizzata e venduta all'ingegner Bozza per pochi soldi. Quel 6 agosto di centocinquantasette anni fa i lavoratori decisero di manifestare fuori la fabbrica e le guardie che furono chiamate spararono sui lavoratori. Manifestarono perché in pochi mesi furono ridotti lavoratori e salari. Il malcontento era così diffuso che, appunto, il 6 agosto del 1863 gli operai decisero di fermare le macchine e suonare la sirena in segno di protesta: una rivolta pacifica, volta a chiedere diritti e garanzie, si trasformò in tragedia. Spararono sugli operai uccidendone quattro: Luigi Fabbricini, Aniello Marino, Domenico Del Grosso, Aniello Olivieri. In base a studi successivi possiamo affermare che ci furono altre vittime, in realtà in ospedale, proprio per le ferite riportate. Quattro uomini, quattro lavoratori napoletani furono uccisi perché provavano a difendere i propri diritti. Per noi la storia non può essere cancellata. Con l'eccidio di Pietrarsa, il 6 agosto è il primo maggio dei lavoratori napoletani. *(Applausi)*.